Onorevoli colleghi, lo scorso 23 giugno si è spento a Roma Stefano Rodotà, insigne giurista, raffinato intellettuale dalla vasta ed eclettica cultura, uomo politico di grande spessore, deputato dalla VIII alla XI legislatura. Nato a Cosenza il 30 maggio 1933 da una famiglia della minoranza linguistica albanese, dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita nel 1955 all'università La Sapienza di Roma, diviene assistente alla cattedra del grande civilista Rosario Nicolò. Nel corso della sua brillante carriera accademica Stefano Rodotà ha insegnato nelle università di Macerata, Genova e Roma, fino a conseguire il titolo di professore emerito di diritto civile. Lunghissimo è anche l'elenco delle università straniere in cui ha esercitato la docenza, in Europa e nel resto del mondo. È stato presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso, responsabile scientifico del Festival del diritto di Piacenza dal 2008, al quale ho avuto il privilegio di partecipare dietro suo invito, ha diretto le riviste giuridiche «Politica del diritto» e «Rivista critica del diritto privato». I suoi maggiori contributi scientifici si concentrano sulla tematica del diritto civile inquadrato in una prospettiva costituzionale, soprattutto con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino, alla protezione della *privacy*, al libero accesso alla conoscenza, sintetizzati nella formula di grande impatto: il diritto di avere diritti. Dopo un'iniziale militanza nel Partito Radicale di Mario Pannunzio, Rodotà viene eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1979 come indipendente nelle liste del Partito Comunista. Rieletto nel 1983, diviene presidente del Gruppo della Sinistra indipendente e fa parte della Commissione parlamentare per le riforme presieduta da Aldo Bozzi. Dopo la svolta della Bolognina, il congresso di Rimini del 1991, aderisce al Partito Democratico della sinistra, di cui sarà il primo presidente del Consiglio nazionale fine al 1992. Eletto Vice Presidente della Camera nella XI legislatura, il 25 maggio 1992 presiede il Parlamento in seduta comune in occasione delle elezioni di Oscar Luigi Scalfaro alla Presidenza della Repubblica. Al termine della legislatura, nel 1994 decide di non ricandidarsi per tornare all'insegnamento universitario. Il suo impegno istituzionale è proseguito anche fuori dalle Aule del Parlamento: primo presidente del Garante per la protezione dei dati personali dal 1997 al 2005; presidente del Gruppo europeo sulla protezione dei dati dal 2000 al 2004; presidente della commissione scientifica dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali nel 2007. Come rappresentante del Governo italiano, ha partecipato ai lavori della Convenzione, guidata dall'ex presidente della Repubblica federale tedesca, Roman Herzog, che nel 2000 predispose la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Rilevante è stato inoltre il suo impegno negli studi sulle prospettive della bioetica, nell'ambito dei quali ha sempre mantenuto un approccio rigorosamente laico incentrato sulla tutela dei diritti di autodeterminazione. In merito ai rapporti tra diritto ed evoluzione del *web*, oltre alla partecipazione all'Internet governance forum dell'ONU, si ricorda il suo contributo nel 2014 come presidente della commissione Internet bill of rights, chiamata a elaborare i principi generali della comunicazione *online* al fine di definire gli indirizzi per le leggi italiane in materia. Un aspetto rilevante della sua ricerca attiene alla protezione della libertà personale nel mondo della rete e dei *big data*, concepiti come spazio neutrale ed egualitario e non come mero strumento di mercato. La carriera accademica e l'impegno politico e istituzionale di Stefano Rodotà risultano fortemente intrecciati al ruolo di intellettuale militante, che lo vede fino all'ultimo protagonista e promotore di numerose iniziative politico‑culturali nonché autore di una copiosa e articolata produzione saggistica. In tutti questi ambiti, la caratteristica del suo stile si è tradotta nella capacità di unire il rigore e la lucidità dell'analisi alla passione argomentativa; il tutto accompagnato da riflessioni giuridiche acute guidate dal faro della tutela dei diritti e della difesa della Costituzione repubblicana. Nel formulare la commossa ed unanime partecipazione del Senato della Repubblica al dolore della famiglia, della moglie Carla e del figlio Carlo presenti in tribuna, degli amici e della comunità scientifica, per la perdita di un grande uomo delle istituzioni, invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.

nel dibattito pubblico Stefano Rodotà è stato spesso definito un costituzionalista. L'appellativo è accademicamente improprio poiché egli è stato un insigne maestro del diritto civile; uno dei massimi della sua generazione per comune consenso. Ma la definizione è probabilmente meno inappropriata se si considera quanto Rodotà abbia saputo calare la Costituzione e i suoi princìpi fondamentali nelle trame dei rapporti interprivati. Non a caso, fu lui a redigere il commento all'articolo 42 della Carta, in tema di proprietà, nel prestigioso «Commentario alla Costituzione» curato da Giuseppe Branca per Zanichelli. In realtà, è proprio la sua capacità di cogliere la valenza costituzionale dei rapporti giuridici tra privati che può aiutarci anche a comprendere il suo percorso politico. Personalmente ho seguito quel percorso fin da quando Rodotà era un giovane e brillante editorialista di «Panorama». Avevo studiato i suoi esordi nell'Unione Goliardica Italiana a quel tempo alcuni dei suoi riferimenti - penso anzitutto a Franco Roccella e Marco Pannella - erano anche i miei. Rodotà era allora il giovane interprete di un nuovo liberalismo, che si proponeva di riempire quel vuoto che aveva portato Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del liberalismo europeo», a definire, forse con eccessiva severità, il liberalismo italiano come una tradizione minore se non assente. In quelle temperie, due correnti del pensiero liberale - quella d'ascendenza francese e giacobina, che si rifaceva ai Lumi, e quella e quella Whig e anglosassone, che si rifaceva alla tradizione inglese e al repubblicanesimo americano - si confondevano e contaminavano vicendevolmente; più avanti si sarebbero divaricate fino al punto di contrapporsi. Un primo bivio si presentò a Stefano Rodotà nel 1979, quando si trovò a scegliere se candidarsi come indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano o in quelle del Partito Radicale. Intraprese la prima strada e, con questa, il tentativo di portare nella tradizione ufficiale della sinistra italiana una ventata di liberalismo che la potesse rinnovare dal punto di vista ideologico. Siamo alla fonte primaria di quel radicalismo di massa che, con il crollo del Muro e la fine del comunismo, si sarebbe candidato all'ideologia ufficiale della sinistra; una sorta di ideologia di sostituzione. Lungo questa via Rodotà si spinse a ritenere che la libertà si sostanziasse in diritti positivi, a loro volta in grado di generare altri diritti, in un'utopica ricerca di autodeterminazione assoluta dell'individuo. Combatté su questo fronte le sue principali battaglie e cercò di rendere questa la divisa identitaria della sinistra dell'Unione europea, di cui egli fu uno dei principali ideatori ed estensori, risponde infatti a questa ideologia, così come anche il suo impegno per la *privacy*, che lo vide promotore dell'*Authority* in Italia, nonché garante europeo. Persino il suo rapporto critico con la sinistra può essere guardato con queste lenti: non a caso, da quella ufficiale si distaccò proprio quando non la vide aderire appieno al suo idealtipo. È evidente che chi concepisce la libertà come imperfezione, legata alle scelte della persona assai più che alle leggi, irrorata dalla tradizione come portato di responsabilità; chi insomma alla scuola francese e continentale ha preferito un liberalismo conservatore di stampo anglosassone; chi individua l'identità europea non nei diritti, ma sulle colline di Roma, Atene e Gerusalemme, ha avuto spesso Stefano Rodotà come avversario e contraddittore. Nondimeno, anche nella contrapposizione - a volte vivace Stefano Rodotà è sempre stato un avversario leale, che ha vissuto la politica come passione e impegno disinteressato e non come calcolo e convenienza. Forse anche per questo, provenendo da una comune radice liberale e dopo averla sviluppata in direzioni addirittura opposte, lo scorso 4 dicembre ci si è ritrovati dalla stessa parte, contro una politica concepita come cinica superficialità. Anche per questo, da avversari, sapere della sua morte è stato un dispiacere autentico e siamo certi che saremo tra quanti - forse anche più di alcuni che erano dalla sua parte - avvertiranno la sua assenza.*(Applausi dai Gruppi PD e*

È stato alla guida di una delle cattedre di diritto civile più rivoluzionarie e innovative e le sue lezioni spaziavano dal diritto di proprietà ai nuovi diritti creati dalle sfide e dalle opportunità offerte anche dalle tecnologie. Ma era sempre molto attento a tutte le problematiche legate alla tutela ambientale. Rodotà è stato un giurista, tecnicamente un civilista e forse non propriamente un costituzionalista, sebbene la sua analisi del diritto non abbia mai mancato di prendere le mosse proprio dalla Costituzione, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che contribuì a scrivere. Furono suoi i primi studi che hanno posto in chiave critica il problema della responsabilità civile. L'individuazione dell'articolo 2043 del codice civile come una clausola generale flessibile per la tutela dei diritti in un mondo che è stato travolto da varie modifiche, anche dal punto di vista giuridico, e dall'introduzione anche di molte tematiche proprio nell'ambito dei diritti. Ha poi aperto la strada ai filoni del danno biologico (e ricordiamo quanto rivoluzionario fu questo principio), del danno esistenziale, nonché della responsabilità oggettiva. È sua anche una lettura che ha posto al centro della riflessione il ruolo delle fonti di integrazione del contratto, spalancando forse anche le porte all'interpretazione di centinaia di forme diverse di contratti atipici Stefano Rodotà verrà dunque ricordato come il giurista delle nuove tecnologie. Le sue proposte si sono poi tradotte in leggi; la legge sul danno ambientale, sulla protezione dei dati personali, nella doppia connotazione europea e nazionale. Forse su molti temi ci troviamo distanti dalle soluzioni che egli proponeva ma non possiamo non apprezzare la finezza delle analisi e dei contenuti delle argomentazioni da lui portate. Di lui, quindi, sicuramente ci resta l'immagine un uomo misurato nei modi, caratterizzato da un intelletto vivace e da una curiosità curiosità infinita. Alla sua famiglia e ai suoi amici esprimiamo il cordoglio di tutto il Gruppo della Lega Nord. Stefano Rodotà è stato una presenza originale nel mondo intellettuale italiano degli ultimi cinquant'anni, perché ha saputo innovare la cultura giuridica del diritto e trasfonderla nell'impegno politico e civile. Di origini cosentine, invece di completare la sua formazione giuridica con il tradizionale viaggio in Germania, privilegia i rapporti con il mondo angloamericano, dove intercetta e da dove importa tra i primi in Italia, con un percorso analogo a quello compiuto da Franco Ferrarotti nella sociologia, la sensibilità per i nuovi diritti; anzitutto diritti civili, intesi nella loro dimensione universalistica di lotta all'oppressione e di tutela della nuda vita, a partire dal convincimento che: «la privazione dei diritti corrisponde sempre alla cancellazione dell'umanità di una persona, che si trasforma in un'ombra destinata prima o poi ad essere cancellata». Proprio diritto civile è la disciplina che insegnerà all'Università di Roma a partire dal 1966, formando generazioni di studenti al rigore del ragionamento, al gusto per il confronto critico, aperto e senza barriere, all'affabulazione e alla enciclopedica erudizione della sua oratoria. Animò anche la rivista «Politica del diritto», con la sua idea del diritto come strumento non di conservazione ma di trasformazione sociale. Di formazione radicale e liberalsocialista, giunse a Roma, scoprì il mondo di Mario Pannunzio, l'UGI, i radicali di Marco Pannella, l'esperienza di comunità di Adriano Olivetti. E a partire dalla sua fondazione a metà degli anni Settanta, iniziò a collaborare con «la Repubblica», con una serie di editoriali puntuali che trasferirono a un pubblico di lettori più vasti il cuore della sua riflessione giuridica, sempre inserita in una sua specifica dimensione politica e civile. Rodotà incontrò la politica, delle istituzioni e nelle istituzioni, nel 1979, quando venne eletto come esponente della sinistra indipendente nelle file, prima del PCI e poi del PDS, di cui sarebbe stato il primo Presidente. E rimase parlamentare per quattro legislature, fino al 1994. Tra i suoi tanti interventi si ricorda quello volto a garantire la permanenza del voto segreto dei parlamentari su questioni relative a diritti sensibili delle persone. Nel marzo 1997 fu eletto presidente dell'organo collegiale del Garante per la protezione dei dati personali, carica mantenuta fino al 2005. Tale funzione gli ha consentito di affrontare - tra le altre cose - il tema della protezione dei dati personali al tempo di Internet e del libero accesso alla conoscenza, sottolineando il bisogno di mantenere il *web* come spazio egualitario, neutrale,

Il primo riguarda il tema della dignità degli «invisibili», del diritto ad avere diritti. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che egli ha contribuito a scrivere per l'Italia, stabilisce in modo vincolante per tutti i Governi che: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Il secondo valore è quello della laicità, intesa non come un contenuto, una sorta di altra confessione, ma come una modalità di pensiero, una componente essenziale - scrive Rodotà - del discorso pubblico in democrazia, uno spazio costituzionale che consente a tutti la convivenza e il confronto.

vanno le condoglianze del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista. Rodotà lascia un grande vuoto; la sua voce e il suo impegno ci mancheranno, ma non la voglia di proseguirne le battaglie nel solco tracciato dal suo esempio. Signor Presidente, ho conosciuto il pensiero e il fascino di Stefano Rodotà, del giurista e dell'uomo politico, per il tramite di amicizie comuni che spesso hanno posto alla mia attenzione la grandezza dell'uomo e la rilevanza dello studioso e, anche se quasi sempre sono stato distante dalle sue posizioni, avendo radici politiche completamente diverse, questo non mi ha impedito di apprezzare molte delle sue teorie e di condividere alcune sue battaglie. In particolare, come amministratore di un paese del Sud ho trovato pienamente convincente la sua posizione giuridica e politica a difesa dei beni comuni. Guardare ai diritti degli utenti, dei cittadini, spesso vuol dire affermare un nuovo concetto di amministrazione pubblica fondato sull'idea che i beni, privati o pubblici che siano, non sempre devono essere oggetto di speculazioni del mercato. Così cercai di fare da sindaco, sottraendo alla vendita uno dei fari più belli delle nostre coste italiane per ricondurlo alla gestione del demanio e del Comune; nello stesso modo, con la mia comunità abbiamo resistito alle speculazioni edilizie nell'area di un bellissimo parco regionale. Le medesime battaglie sono state condotte con il supporto di Stefano Rodotà per il vicino teatro Valle, quindi il tema dei beni comuni si affermava ovunque. Un altro suo impegno da me condiviso è stato quello a difesa della vigente Costituzione in occasione del *referendum* del 4 dicembre scorso, come è stato ricordato anche negli interventi precedenti. Magari i punti di partenza erano molto diversi, ma per chi come noi si è impegnato a difesa delle ragioni del no trovare un autorevole compagno di viaggio come Stefano Rodotà non è stato certo insignificante. Contrapporsi all'arroganza delle posizioni del sì con gli anticorpi e con la *scientia iuris* di valenti accademici come Rodotà ha reso molto più facile il nostro compito. Ancora, da posizioni politiche ed ideologiche diversissime ho avuto modo di apprezzare quanto affermato nel suo volume «La vita e le regole». Nell'*incipit* troviamo scritto: «Può il diritto, la regola giuridica, invadere i mondi vitali, impadronirsi della nuda vita, pretendere che il mondo debba "evadere "evadere dalla vita"?». Viviamo «in una società strapiena di diritto, di regole giuridiche dalle provenienze più diverse, imposte da poteri pubblici o da potenze private, con un'intensità che fa pensare, più che ad una necessità,

Questi concetti oggi sono di grandissima attualità e dovrebbero essere oggetto di continue riflessioni da parte di tutti noi. Esprimo quindi in questa sede la partecipazione al cordoglio dei familiari

Signor Presidente, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Stefano Rodotà sette anni fa. L'ho conosciuto da operaio metalmeccanico e delegato FIOM della FIAT di Melfi. Sono rimasto subito colpito dal fatto che per lui «diritto» non era una parola astratta ma una realtà da difendere giorno per giorno. Parlava di diritto ad avere una famiglia normale per gli omosessuali, di diritto alla *privacy*, di cui è stato garante dal 2000 al 2004, di diritto ad una morte dignitosa, di diritti dei lavoratori; insomma l'esatto contrario, dobbiamo dirlo, di quello che a volte succede in queste Aule, dove i diritti sono a seconda di chi o cosa. Sei sempre stato coerentemente dalla parte giusta, e io aggiungo anche dalla parte dei deboli, quando quasi tutti erano affascinati dal potere economico padronale e per questo si cercava in tutti i modi di giustificare il *referendum* di Pomigliano. Come ricorderete, in cambio di lavoro gli operai dovevano rinunciare ai propri diritti - lo ricordate?

Tu, Stefano, dicevi che Marchionne non nasce dal nulla; Marchionne nasce da decenni nel corso dei quali diritti, legalità e magistratura sono stati oggetto di un violento attacco diventava chiaro nelle sue idee). Avevi visto giusto; Pomigliano doveva essere un'eccezione, lo ricordiamo tutti, e poi è diventato una regola: la regola, Presidente. Oggi vediamo ciò che accade nel mondo del lavoro dove gli operai vengono licenziati e non si può muovere nessuna critica al padrone, pena querele. Bisogna solo dire grazie a Stefano Rodotà che, a volte in un panorama di pochezza politica e a volte anche di un vuoto di democrazia, non solo non ci ha mai abbandonati non ci ha mai abbandonati ma ha condotto insieme agli operai e agli ultimi una battaglia vera di civiltà. «La privazione dei diritti corrisponde alla cancellazione dell'umanità», dicevi, e ti sei battuto fino all'ultimo per questo. Senza nulla togliere a nessuno, se fosse stato possibile il voto operaio, saresti stato orgogliosamente il nostro presidente. Ma, si sa, agli operai è anche vietato votare i propri rappresentanti, e questa è la realtà. Sì, caro Stefano, sei stato un vero professorone, di quelli che hanno fatto la storia di questo Paese e per questo sarai ricordato e, come tutti i grandi, ci hai lasciato un ultimo regalo: sei stato in prima fila a difendere la nostra Costituzione, che per noi è sempre la più bella. Grazie Stefano, ci mancherai davvero tanto. Noi di Sinistra Italiana continueremo la tua, la nostra battaglia e, come tu hai scritto, continueremo a pretendere il diritto di avere diritti per tutti, nessuno escluso. Ciao professore, sì, hai ragione anche sul fatto che siamo obbligati alla civiltà se vogliamo una democrazia degna di questo Paese. Sinistra Italiana abbraccia con tutto il cuore i suoi familiari che sono presenti oggi Signor Presidente, Stefano Rodotà può essere ricordato in molti modi: come intellettuale, come esimio docente di diritto, il cui impegno accademico si è sempre intrecciato con quello politico, come parlamentare e primo autorevole garante della *privacy*. Certamente è stato un protagonista della vita civile e politica del nostro Paese. Ma accanto a questo, ci piacerebbe ricordarlo innanzitutto per il privilegio che il Movimento 5 Stelle ha avuto nel condividere con lui la battaglia in difesa della nostra Costituzione,

In quell'occasione, Rodotà ebbe modo di dire che il tentativo di impadronirsi della Costituzione, condotto con determinazione ed aggressività, era fallito chi aveva cercato di impadronirsi della Costituzione aveva ottenuto il risultato opposto, quello cioè di richiamare l'attenzione di tutti i cittadini sull'importanza della Costituzione stessa. Ma soprattutto vogliamo ricordare Stefano Rodotà per l'onore che quattro anni fa concesse al Movimento 5 Stelle accettando la candidatura a Presidente della Repubblica. In quei giorni del 2013, giorni che non dimenticheremo, Rodotà non è stato semplicemente il candidato alla Presidenza della Repubblica del Movimento 5 Stelle: Rodotà divenne il candidato di tutta quella parte del Paese che si riconosceva nella sua storia, nei suoi valori, nelle sue battaglie per i diritti. La scelta di proporlo per il ruolo di Presidente venne presa dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Quella di sbarrargli la strada, invece, fu la decisione dei parlamentari dei vertici del PD, che oggi hanno la responsabilità di non aver voluto al Colle un uomo perbene e soprattutto innamorato della nostra Costituzione. In tanti, non solo nel Movimento 5 Stelle, ci siamo chiesti come sarebbe cambiata l'Italia se le cose fossero andate diversamente e Stefano Rodotà fosse salito al Quirinale. Avremmo oggi probabilmente un'Italia più libera e più giusta, più onesta e più solidale. Certamente con la sua scomparsa siamo tutti un po' più indifesi, più fragili e più soli. Grazie presidente Rodotà, noi abbiamo provato a darti il riconoscimento che meritavi, e probabilmente è proprio questo Parlamento che non ti meritava. ricordo con rispetto e commozione Stefano Rodotà, la sua profonda cultura, la sua sincera passione sociale e politica, la sua coerenza. Vedendo il *curriculum*, colpisce il fatto che negli ultimi anni della sua vita si sia dedicato ed abbia messo a disposizione la sua cultura giuridica in un soggetto completamente nuovo, del quale sono protagonisti soprattutto i giovani e cioè il nuovo sistema informatico, le questioni *online* e la *privacy* collegata a questo Stefano Rodotà è stato un intransigente avversario politico di Forza Italia ed ha più volte espresso giudizi assai severi nei confronti del nostro *leader* Silvio Berlusconi, severità resa ancora più evidente dalla sobrietà ed asciuttezza del suo eloquio, dalla mitezza del suo sguardo. La regola della democrazia ha fatto sì che ci si sia trovati schierati dalla stessa parte nella sua ultima battaglia politica, il *referendum* costituzionale. Con rispetto e commozione, rendo omaggio alla sua memoria e saluto la moglie ed il figlio.

Democratico. La prassi del Senato prevede la commemorazione in Aula della scomparsa dei nostri colleghi senatori ed è molto raro che lo si faccia per personalità che non hanno mai seduto su questi banchi. Se oggi commemoriamo Stefano Rodotà, lo facciamo perché sentiamo di dover onorare un grande italiano, nei cui confronti anche chi non ha sempre condiviso le sue posizioni sa di avere un debito per la coerenza e la forza del suo pensiero e per la lealtà dei suoi comportamenti. In un tempo nel quale la fermezza delle idee non è certo la caratteristica più rilevante del nostro costume nazionale, anche solo queste doti sarebbero sufficienti per un pubblica riconoscimento da parte del Senato. Ma Stefano Rodotà non è stato solo coerente con i suoi principi e leale con gli interesse del Paese. È stato molto di più. Ha combattuto importanti battaglie civili, istituzionali e politiche ed è stato professore, parlamentare, editorialista e saggista e in tutto quel che ha fatto ha sempre eccelso per una dote su tutte: il rigore morale delle sue posizioni e la visione larga e profonda con la quale ha saputo trattare ogni questione che ha voluto o gli è capitato di affrontare. un suo vecchio amico, ricordandolo, ha sottolineato come questa sua ansia di cogliere la complessità dei fenomeni del suo tempo fosse visibile sin dall'inizio della sua vita di studioso. I suoi primi lavori civilistici sul contratto, sulla responsabilità e sulla proprietà, si imposero immediatamente all'attenzione della comunità accademica e non solo per la novità delle intuizioni scientifiche, ma anche per la straordinaria capacità di mettere in rapporto i più rilevanti istituti del nostro dritto civile con i principi fondamentali della Costituzione e con le fondamenta del nostro diritto pubblico. Rodotà con grande laicità ha fatto vivere la Costituzione nei fatti della nostra vita quotidiana. In questi giorni, subito dopo la sua scomparsa, Stefano Rodotà ha ricevuto tanti riconoscimenti da parte di chi ha condiviso le sue posizioni e anche da chi aveva opinioni diverse. Questo è un segno, inusuale, di vero rispetto e di sincera considerazione. Chi ha scritto o parlato di lui, senza eccezione alcuna, ha messo in rilievo la sua straordinaria capacità di non limitarsi mai a esaminare i problemi da affrontare solo nel loro ambito specialistico, ma di considerarli sempre nel nel loro contesto storico, istituzionale, culturale, sociale e giuridico. Questo suo metodo lo ha sempre aiutato ad andare al fondo dei problemi, a meglio comprenderli e a meglio farli comprendere. È una qualità che ha ingigantito le sue analisi, sia scientifiche che politiche. Sostenitore instancabile delle libertà civili e dei diritti di ogni singolo cittadino, non perdeva mai di vista gli interessi generali della società nel suo complesso. Grande appassionato delle istituzioni nazionali ed europee, sapeva collegarne l'evoluzione ai mutamenti nei rapporti economici e sociali. Maestro del diritto civile italiano conosceva in profondità gli ordinamenti giuridici di gran parte delle democrazie occidentali. Fermo sostenitore del diritto alla *privacy* e della necessità di una sua rigorosa tutela, ha sempre difeso la libera stampa e il diritto dei cittadini a essere informati con quanta maggiore profondità possibile. In una parola, Stefano Rodotà aveva compreso la straordinaria complessità dei problemi del nostro Paese. Conosceva i nostri ritardi e le nostre contraddizioni e ha messo la sua competenza di luminare del diritto e la sua sensibilità politica di uomo della sinistra italiana ed europea al servizio della realtà del suo tempo. Nel farlo non si è mai risparmiato nella battaglia politica, sempre però combattendo nel merito dei problemi e mai per pregiudizio. In termini politici, possiamo anche dire che Stefano Rodotà, talvolta sostenendo gli interventi che approvava, altre opponendosi a riforme che non condivideva, ha speso una parte ampia della sua vita nel tentativo di sciogliere le corpose contraddizioni di una società in tumultuosa trasformazione, dove non è semplice trovare un equilibrio tra l'interesse generale e i diritti individuali, tra le regole del mercato e la giustizia sociale, tra la riservatezza di ciascuno di noi e la bulimia informativa dalla quale siamo sommersi fino al collo. Concludo ricordando con molta personale amicizia un aspetto della personalità di Stefano Rodotà che mi ha sempre molto colpito. L'ho ascoltato un'infinità di volte in dibattiti pubblici sulle grandi questioni politico-istituzionali, sulle libertà e sui diritti civili, tutti temi che l'hanno visto fortemente impegnato negli ultimi decenni. E mi è anche capitato con una qualche frequenza di discutere con lui nelle più svariate occasioni. In privato Stefano Rodotà era un conversatore molto brillante e nei dibattiti pubblici era straordinario nel tenere testa a chiunque sostenesse idee diverse dalle sue. Lo aiutavano la sua padronanza assoluta del diritto e la sua sensibilità politica, ma anche una vastissima cultura economica, letteraria, musicale, storica e financo la conoscenza profonda delle nuove tecnologie, di cui aveva avvertito con grande anticipo le potenzialità positive in termini di progresso della società, ma anche le insidie e i pericoli che ne potevano derivare per i diritti delle persone. In tutte queste occasioni ho sempre visto Stefano Rodotà difendere le sue posizioni non solo con ricchezza argomentativa, ma anche con una fermezza e un'intransigenza che gli venivano da convinzioni profonde e radicate. Ebbene, anche nei dibattiti più combattuti, nelle conversazioni più accese, anche quando lui ed io sostenevamo posizioni diverse o vedevamo le cose da diversi punti di vista, non l'ho mai visto perdere la mitezza che lo contraddistingueva, mai visto sue reazioni scomposte, mai percepito che per battere dialetticamente l'avversario fosse tentato dall'abbandonare il filo della logica e la compostezza del ragionamento. Abbiamo tutti molto da ricordare e da imparare dalla memoria di Stefano Rodotà. A noi che tutti i giorni affrontiamo lo scontro politico nell'Aula e nelle Commissioni del Senato, può essere prezioso ricordarlo mentre combatteva le sue battaglie politiche o culturali senza mai insultare l'avversario e senza mai aggredirlo. Vinceva sempre con la forza della sua cultura e dei suoi argomenti.

alla famiglia, alla signora Carla, al figlio Carlo e alla figlia Maria Laura, e per precisare che Stefano Rodotà era innanzitutto un giurista, come è stato ripetuto più volte in quest'Aula. Non di meno diritto, ma di miglior diritto sentiva l'esigenza e la sentiva con una capacità di precorrere i tempi che certamente in qualche momento era addirittura apparsa visionaria. Discute in questi giorni il Senato della Repubblica di un disegno di legge che riguarda il diritto all'identità dei bambini, con l'imposizione del nome del padre e della madre; mi diede l'onore di aprire una lezione al suo corso di diritto privato alla Sapienza esattamente su questo tema più di vent'anni fa. Non era visionarietà, era piuttosto questa concezione del diritto come modello, strumento da mettere in mano a un'umanità che di quello aveva bisogno, anche se ancora quel bisogno non era stato espresso, sistematizzato, compiutamente addirittura accettato dalla società italiana. Così è stato per i temi che sono stati qui ricordati, ma io voglio ricordare innanzitutto il tema del diritto all'uguaglianza, o meglio del diritto alle pari opportunità per soggetti che si trovino in condizioni di differenza. Era un giurista che ha sempre pensato che essere giurista dovesse avere un'utilità. Ricordo che accettò un mio commento a un suo libro «Repertorio di fine secolo», uno dei suoi libri secondo me più interessanti e più utili; era un giudizio di utilità di quel libro e lui mi disse che, per un giurista, essere utile è il più grande dei riconoscimenti.

poche figure, che fino a questo momento hanno assistito il Paese, di intellettuale e insieme politico, cioè di chi riesce a rendere il proprio esercizio della politica e anche la propria scelta di campo, scelta competente, informata, lungimirante, ordinante il pensiero e il dibattito pubblico. Ovviamente, quando scompare un uomo della sua personalità e - usiamo questa parola - del suo carisma molti di noi si sentono epigoni ed è giusto che sia così e credo sia anche di consolazione e conforto per la sua famiglia. Ma è importante essere in grado di cogliere che questo carisma, questa capacità ordinante del dibattito pubblico, anche intorno a temi controversi, a temi di frontiera, era il frutto di una conoscenza che è la conoscenza umana, ed era la molteplicità delle conoscenze che ne facevano appunto un intellettuale di primissima qualità. Scompare Stefano Rodotà, scompare dunque una di queste rare figure e, per quanto mi riguarda, scompare anche un amico.

n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*** nella seduta pomeridiana del 21 giugno sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà. Presidente, colleghi, in questi giorni, in queste ore, mentre noi stiamo discutendo in Parlamento la modifica del codice antimafia, le organizzazioni criminali continuano a fare il loro mestiere e a radicare il loro potere economico e finanziario sulla piazza globale, non soltanto europea. Stanno privilegiando i Paesi della nuova Europa, ancora in via di sviluppo e destinatari di ingenti risorse comunitarie destinate, in prevalenza, alla realizzazione di infrastrutture primarie. Lo stanno facendo in Romania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia. Ce lo dicono numerosi indicatori: dalla mobilità delle imprese, anche in odor di mafia, agli atti d'indagine, anche di questi giorni, su ditte specializzate nell'edilizia, nel manifatturiero, nella ristorazione, nel gioco e nel divertimento. A conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, che le organizzazioni criminali hanno dismesso da tempo le vesti della mala esclusivamente violenta preferendo indossare quelle più comode e anonime dei *broker* e degli imprenditori, allargando la propria sfera d'influenza, allontanandola dai centri investigativi italiani capaci, più di altri, di riconoscerle e colpirle - e spostandola lì dove ancora resiste la comoda convinzione che mafia, camorra e 'ndrangheta siano patologie tutte italiane. Pian piano i Paesi europei stanno adeguando la propria legislazione, senza però comprendere fino in fondo la pervasività di quelle organizzazioni, capaci di inquinare economia e politica senza armi convenzionali, ma con la corruzione. Ma è proprio dall'Europa che certamente può arrivare la spinta trainante per il futuro contrasto alle mafie, spinta che necessita di una capacità di analisi europea, se non globale, dei mezzi di contrasto alle organizzazioni mafiose, appunto dalle misure di prevenzione e dalla confisca dei beni. E sono proprio questi i punti fondamentali del provvedimento al nostro esame: dalle forme del procedimento di prevenzione alla disciplina della gestione e della destinazione dei beni confiscati. Si è provveduto infatti a incrementare le tipologie di soggetti pericolosi e quindi passibili di essere sottoposti a misure di prevenzione: oltre agli indiziati di mafia, ci sono coloro che hanno dato assistenza agli associati, ma anche gli indiziati dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, elevati a categoria a pericolosità qualificata, al pari degli indiziati di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso. A voler rimarcare, dunque, anche la pervasività dei sistemi corruttivi, capaci di modificare profondamente non soltanto l'andamento della pubblica amministrazione e, più in generale, del sistema Stato, ma anche il rapporto tra questi e i cittadini. Lo aveva ricordato nelle ultime settimane il capo della procura di Roma, Giuseppe Pignatone, citando la Cassazione a proposito di Mafia Capitale: «Nella sua storia, la criminalità organizzata - aveva detto ha sempre fatto ricorso alla corruzione, fermo restando che mafia e corruzione sono due realtà diverse e non sempre dove c'è l'una c'è anche l'altra. L'elemento di novità è che la corruzione è diventata strumento e manifestazione dell'intimidazione mafiosa». L'attività corruttiva viene scelta innanzitutto perché gli atti violenti allarmano l'opinione pubblica e attirano l'attenzione di polizia e magistratura; inoltre, la mescolanza tra il mondo mafioso e quello "altro" "altro" genera influenze reciproche, così che le mafie accettano le regole, a volte mutuano persino il linguaggio, dei loro interlocutori. I criminali, infine, stanno bene attenti a non mettere in difficoltà con episodi violenti l'amministratore o il funzionario amico, perché questi possa aggiustare la gara d'appalto con i suoi metodi e i suoi tempi. È in questo contesto, dunque, che vanno lette le singole riforme contenute nel codice antimafia. Particolare rilievo ricopre, per esempio, la proposta, già fatta dal Governo con l'Atto Senato 1647, di un ulteriore potenziamento dell'istituto della cosiddetta confisca allargata, di cui all'articolo 12-*sexies*. Nell'ottica di estendere la sua sfera di operatività, si prevede l'espresso richiamo ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di rito, nel cui elenco sono stati inseriti molto opportunamente i più gravi delitti ambientali (di disastro e di inquinamento) e il delitto di traffico organizzato di rifiuti. Il testo ora in esame si muove nella direzione della valorizzazione delle affinità della confisca allargata con la confisca di prevenzione, con il chiaro intento di affinare un armamentario giuridico con indiscutibili profili di complementarietà: in questa prospettiva, per esempio, la legittima provenienza dei beni non potrà più essere giustificata dal proposto adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale (in questi termini, per la confisca di prevenzione, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite). La riforma, dunque, cristallizza in norma ciò che sinora è solo un'indicazione giurisprudenziale, sia pur qualificata. Come la confisca di prevenzione prescinde, per sua struttura, da un accertamento di responsabilità per i delitti la cui commissione costituisce lo sfondo in cui essa si inserisce, così la confisca allargata si affranca, nei limiti del possibile, dalle sorti del procedimento penale, per soddisfare al meglio l'esigenza,

rendendo applicabile alla confisca allargata la disciplina della confisca di prevenzione, comprese le regole relative alla tutela dei terzi e all'esecuzione del sequestro. In questa dimensione generale, va considerato anche l'interesse riservato al profilo della specializzazione delle sezioni di tribunale che trattano la materia della prevenzione: una per distretto, conservando l'eccezione dei circondari di Trapani e Santa Maria Capua Vetere. Bene sarebbe stato, però, preservare la *ratio* ermeneutica delle due eccezioni, precedenti alla nuova geografia giudiziaria, allargandole ai tribunali di Marsala e Napoli Nord, competenti a decidere sulla cosca che fa capo a Matteo Messina Denaro e ai maggiori e più strutturati *clan* della camorra napoletana e casertana, attualmente nella disponibilità - si fa per dire - dei tribunali di Napoli Nord. L'esigenza di specializzazione in un settore di obiettiva complessità e delicatezza appare indubbia, anche tenendo conto, da un lato, dell'incremento della qualità e quantità dei procedimenti di prevenzione e, dall'altro lato, dell'esigenza di uniforme applicazione di una generale istanza di garanzia della trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Nessun progresso sul versante dell'efficienza può dirsi, infatti, stabilmente conseguito se non accompagnato da un corrispondente adeguamento dei meccanismi di tutela dell'effettività delle garanzie difensive e dei diritti dei terzi in buona fede. Vanno, dunque, apprezzati gli sforzi riformatori volti a far conoscere alle parti,

e a rendere maggiormente efficace il procedimento di prevenzione patrimoniale e l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Si propongono innovazioni rivolte all'obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali. Soprattutto, con l'articolo 34-*bis* si introduce l'istituto del controllo giudiziario in applicazione sostitutiva della amministrazione giudiziaria, nei casi in cui l'agevolazione dell'attività di soggetti sottoposti a misure di prevenzione non assuma carattere di stabilità e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività di impresa. È il caso, per esempio, delle aziende che un tempo erano colpite dalle cosiddette informative atipiche, spesso perché i titolari delle stesse avevano subito estorsioni non denunciate o perché nei passaggi di cantiere avevano assorbito manodopera contigua ai *clan*. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa e introduce un intervento meno invasivo di vigilanza prescrittiva affidata a un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Agli interventi fin qui indicati si accompagnano alcune modifiche - non più rinviabili, dopo la scoperta di comportamenti illeciti in alcune sedi giudiziarie -finalizzate a rendere maggiormente trasparenti i criteri di nomina degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, in modo da assicurare la rotazione degli incarichi e la corrispondenza tra profilo professionale dell'ausiliario e tipologia dei beni appresi in sede preventiva. La linea di intervento che riguarda la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un capitolo fondamentale in una rinnovata strategia di aggressione all'accumulazione illecita di capitali. È emersa, inoltre, una visione dell'Agenzia nazionale come struttura con funzioni di ausilio al giudice delegato, dal momento del sequestro e fino alla confisca di secondo grado. Ad essa è attribuita l'amministrazione e la destinazione dei beni dopo l'esaurimento del giudizio di merito. Il ruolo dell'Agenzia in fase di sequestro è orientato ad agevolare l'assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende agli enti territoriali o del terzo settore per finalità istituzionali o sociali. In questo senso, è apprezzabile l'esigenza di orientare la prospettiva in funzione di una «redditività» dei beni, non tanto in senso strettamente economico, ma di più ampio respiro, da intendersi come affermazione della legalità e della presenza dello Stato come risposta ai bisogni sociali della collettività. La valorizzazione dei beni confiscati costituisce un punto essenziale della riforma nella prospettiva di contemperare le esigenze della giurisdizione con le esigenze operative della gestione dei beni fin dal sequestro. L'obbiettivo non è solo quello di rafforzare la capacità di gestione dinamica dei beni nella fase giudiziaria tramite l'assegnazione, come visto, di risorse professionali adeguate, cui attingere per la nomina degli amministratori, ma anche di definire gli strumenti di programmazione e attuazione delle politiche di riutilizzo in termini di *welfare* e inclusione sociale, di promozione cooperativa e di imprenditorialità giovanile, di tutela del lavoro e di nuova occupazione, di sviluppo economico e produttivo. Per i beni confiscati si consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Un passo avanti che va nella direzione da tempo auspicata dagli amministratori locali, superando, senza pregiudizio, il non sempre sostenibile obbligo del riuso di immobili non idonei e fatiscenti, il cui impiego imporrebbe costosissimi lavori di adeguamento statico, antisismico e antincendio. In altre parole, un ulteriore costo per la collettività.

che non intenda collaborare con determinazione all'approvazione di norme che vadano nella direzione del contrasto alla criminalità organizzata. Credo non vi sia

approvati dai vari Governi che si sono succeduti. Ricordo anche - e perché no? - incisivamente i Governi presieduti dal presidente Berlusconi. Quindi, la lotta alla criminalità organizzata è stata sempre una battaglia sostenuta da tutte le forze politiche del nostro Paese.

votato favorevolmente da alcune forze politiche e contrastato invece da altre forze presenti in Aula. questo perché un eventuale voto contrario si presta alle più ambigue interpretazioni. Pare quasi che si vogliano fare sconti alla criminalità organizzata; che non si voglia collaborare nella lotta alla criminalità. come in Commissione il senatore Caliendo e il relatore Lumia hanno dato spunti correttivi al provvedimento, accolti anche dal relatore Pagliari - è stato in qualche modo corretto qualche errore che pur vi era nella stesura che ci proveniva dalla Camera - a un certo punto, non si sa perché, questi rilievi, forse ancora più corretti e più giusti, non sono stati recepiti. Mi si dice che non sono stati presentati emendamenti:

rigettano, le forze politiche devono correggere di intesa. E qual è il *vulnus* che preoccupa chi allo stato deve dire no a questo provvedimento? Il *vulnus* è rappresentato dall'equiparazione dei reati contro la pubblica amministrazione ai reati di mafia.

È chiaro che non ci può essere questa equiparazione e diventa paradossale quando non ci si rende conto che, ad esempio, per il reato di peculato d'uso, si prevede la possibilità di avviare le procedure di prevenzione. Ricordo che il reato di peculato d'uso commesso dal pubblico amministratore che utilizza un foglio di carta, un telefono o un'auto di servizio per fini personali.

quanto sia più odioso e di allarme sociale il reato di femminicidio.

dovremmo ritenere applicabili le misure di prevenzione per tutti i reati. Per quanto mi riguarda, i reati sono tutti odiosi, ma quelli per i quali si attiva una procedura di prevenzione devono essere necessariamente di elevata pericolosità sociale e non credo

Varie sono state le pressioni giunte da soggetti esterni al Parlamento. Io personalmente ho espresso ammirazione e apprezzamento per chi, esterno al Parlamento, ha ha speso il suo tempo e impegnato parole e voce per sollecitare una convergenza tra forze politiche che su questo punto erano in discordia. ieri ho partecipato a un convegno insieme a don Luigi Ciotti, esterno al Parlamento, che in pubblico ha ha affermato la necessità di equiparare i reati contro la pubblica amministrazione ai reati di mafia.

in modo che questo Parlamento, questo Senato, approvi a larghissima maggioranza un provvedimento di tale delicatezza. Ed è qui la delicata funzione del relatore. Il relatore deve percepire questi

Mi permettevo, dalla modestia della mia preparazione, di sollecitare quantomeno un collegamento con l'articolo 416 Il reato contro la pubblica amministrazione, la corruzione, il peculato sono reati odiosi ma possono divenire di allarme sociale solo quando sono commessi in forma associativa, e quindi come associazione a delinquere. si risolve la preoccupazione di un cittadino che ha commesso un delitto, per quanto sanzionabile ma di lieve entità, quale può essere un peculato d'uso, e, contemporaneamente, si soddisfa quella esigenza gridata dalla dottrina italiana, dai giuristi del nostro Paese che hanno lanciato l'allarme per un provvedimento di questo genere. Io voglio votare un provvedimento che contrasti la criminalità organizzata. E voi mi dovete porre nelle condizioni di poterlo votare. Voi non mi potete fare il torto (mi riferisco alla maggioranza maggioranza di Governo) di non votare un provvedimento che va a contrastare la criminalità organizzata. Voi mi ponete in una condizione di disagio di coscienza nel dover dire no. Ed è quindi questo mio un grido: correggetelo! Correggete questi punti. Poi c'è il problema anticipato

circondariale antimafia a Santa Maria Capua Vetere e non a Napoli Nord, ancorché i territori di maggior frequentazione malavitosa fossero di competenza del tribunale. Se questo volete farlo, fatelo. Non mi appassiona più di tanto. Così come non mi appassiona la riforma, che anzi forse condivido, sulle agenzie, spostando la sede da Reggio Calabria a Roma e creando altre sedi sul territorio nazionale. Allo stesso modo accolgo con favore la possibilità di vendere i patrimoni confiscati e non dati in uso talvolta a chi ne fa un cattivo uso. Lo Stato fa cassa, ed ha bisogno di fare cassa, ma correggete il punto centrale di questo provvedimento, questa scellerata equiparazione che non trova conforto né nel diritto né nella dottrina né nel Paese. Fate questo e noi non avremo problemi a votare il provvedimento e voi potrete essere orgogliosi per aver fatto votare questo provvedimento dalla maggioranza del Senato. Non ve ne andate come guitti sotto al muro con il provvedimento in tasca. Non fa bene a voi, non fa bene a noi, non fa bene al Paese. Vi prego, correggetelo. E all'esito delle vostre determinazioni il mio Gruppo assumerà la decisione se votare a favore o meno.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia è sempre stata pronta ad approvare leggi volte a favorire e rendere più efficace la lotta contro la criminalità organizzata, contro le mafie e, quando ha avuto responsabilità di Governo, ha portato avanti una guerra senza quartiere alle organizzazioni criminali cogliendo anche numerosi successi.

Pertanto, anche in questa occasione abbiamo lavorato e intendiamo continuare a farlo perché il provvedimento in esame sia il più efficace possibile

La lotta alla criminalità organizzata può e deve essere condotta anche con strumenti particolari che in altri settori non potremmo introdurre, perché potrebbero essere in contrasto contrasto con la Costituzione o anche con documenti di diritto internazionale. La questione della criminalità mafiosa e della criminalità organizzata può e deve essere condotta con mezzi straordinari che incidano in modo efficace nella realtà e possano portare alla sconfitta e quantomeno a un efficace perseguimento di questo fenomeno.

quelle che in medicina si definiscono le metastasi, che si sono manifestate anche ben lontano dai luoghi dove tradizionalmente si è abituati a immaginare la presenza di questo fenomeno, questo fenomeno, che crea danni diretti in tutti i casi in cui incide in modo fortemente negativo su determinate realtà locali.

è attiva spesso ci si trova di fronte a una fuga delle attività economiche o anche delle singole persone che, non

perché temono, o addirittura hanno sperimentato, la realtà dei taglieggiamenti, delle infiltrazioni, a volte anche nella pubblica amministrazione e in tutti gli organi dello Stato (nella politica, ma non solo), e pertanto cancellano la possibilità di una crescita economica e dunque le speranze e il benessere di molte persone. ancora dell'altro: non soltanto il danno all'insieme della realtà economica di tante parti del Paese, ma anche un danno all'immagine complessiva del Paese, Pertanto non possiamo mostrare debolezza nella lotta al crimine organizzato e dobbiamo essere pronti ad esaminare, come dicevo, tutte le norme che possono essere d'aiuto in questa lotta.

esageratamente severe che indicano molto spesso un insuccesso nell'applicare le leggi normali, quindi un insuccesso di carattere generale. Manzoni ce ne fornisce un esempio citando le famose gride,

effettuavano soprusi vari ai danni di altre persone, imponevano determinate realtà, impedivano matrimoni (e questo si attagliava al romanzo)

Queste ulteriori gride, ci dice Manzoni, si estendevano non soltanto a chi aveva fama di essere uno di questi malviventi, uno di questi bravi, ma anche a coloro che vestivano

In tal modo venivano criminalizzati comportamenti che, di per sé, non costituivano alcun crimine (avere i capelli lunghi non è pericoloso per nessuno, al limite per chi li porta se gli vanno davvero negli occhi) solo per far vedere che si facevano le cose sul serio. In In questo caso, nel provvedimento in esame ci sono delle parti che lasciano quantomeno perplessi. All'articolo 1 si propone di estendere alcune misure cautelari,

dal senatore che mi ha preceduto, tutti i reati, se le leggi sono scritte bene, sono odiosi, per cui si dovrebbe applicare qualunque misura a qualunque reato, può andare bene dal punto di vista filosofico e non dal punto di vista pratico e neanche dal punto di vista del rispetto del diritto: ci devono essere risposte proporzionate alla gravità

con il pericolo che persone alle quali ben si attaglierebbero queste norme speciali o emergenziali possano poi invocarne l'incostituzionalità. E sarebbe davvero paradossale subire una sconfitta non già sul campo, dove non sempre le azioni di indagine, di arresto e di contrasto alla criminalità possono avere successo (in tutte le guerre è impossibile vincere su ogni singolo confronto), ma davanti alla Corte costituzionale. Questo sì sarebbe un danno pesantissimo per il nostro Paese: una norma contro la mafia bocciata dalla Corte costituzionale.

la pistola nel piatto di spaghetti e altre allusioni di questo genere). Noi non abbiamo bisogno di queste cose. Noi abbiamo bisogno certamente di una lotta efficace, di norme che rispondano alle esigenze delle indagini, ma abbiamo anche bisogno di non dimostrarci deboli ed inefficaci, perché oggi non è debole e inefficace la lotta alla criminalità organizzata, per cui non dobbiamo approvare norme che somiglino alle gride, quelle certamente inefficaci, eccessive e velleitarie dell'Italia del Cinquecento e del Seicento descritta dal Manzoni, perché otterremmo l'effetto opposto. Credo che ben altri siano gli strumenti che devono essere usati per dare il messaggio chiaro che si è contro ogni tipo di illegalità, e questo deve venire dai massimi vertici del Paese, a cominciare naturalmente dal Parlamento, dal Governo e da tutte le strutture della pubblica amministrazione. Non dobbiamo arrivare a citare il fatto che il Governo non metta in atto una sentenza della Corte costituzionale, magari riguardante le pensioni. Non dobbiamo arrivare a citare il fatto che che certe norme, che impongono di indire gare di appalto per determinati settori della nostra economia, poi vengano apertamente aggirate. Dobbiamo fare esattamente il contrario, ossia cercare di porre rimedio

dagli atti compiuti dai massimi organi istituzionali del nostro Paese, si percorra sempre il solco della più rigorosa ed efficace legalità.

di criminalità organizzata, indubbiamente possono esserlo, e quindi estendere determinate misure preventive a tali casi può avere una sua giustificazione. Ma

non meritano e non conserveranno né l'una, né l'altra. Per cui attenzione: sacrificando la libertà in nome della sicurezza, si finisce per non fare sicurezza e intanto e intanto si perde un pezzo di libertà. Sono convinto che tutte le parti politiche rappresentate in quest'Assemblea abbiano la volontà di rispettare la nostra Costituzione, rispettare e far rispettare la legge la legge e i diritti dei cittadini, i quali sono - come dice la Costituzione - innocenti fino a che non viene dimostrato il contrario. Per quanto riguarda le norme nei confronti degli indiziati (e la parola «indiziati» ricorre diverse volte

cerchiamo di scrivere norme che distinguano chiaramente lo Stato e la legalità. La Costituzione è la fonte della nostra legalità. Chi è fuori dalla legalità deve essere combattuto, ma dobbiamo farlo con le armi del diritto e della nostra Costituzione.

dopo circa tre anni da quando in quest'Aula abbiamo votato la risoluzione della Commissione antimafia con cui si chiedeva una riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, finalmente siamo all'atto finale per dare seguito a quella volontà. Il disegno di legge che siamo chiamati ad approvare, infatti, seppur partito dalla Camera su iniziativa parlamentare, è figlio di quella relazione. L'articolato modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e riforma l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, per migliorarne l'operato nella gestione e dismissione dei beni, ma non solo. Come già altri prima di me hanno evidenziato, è un intervento che viene chiesto da anni da chi, sul terreno del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ha chiaro che per colpire al cuore le mafie è necessario che l'aggressione ai patrimoni illeciti che ne sono il frutto sia effettiva.

cioè come un tutt'uno, sia nella fase dell'aggressione vera e propria - sequestro e confisca in cui lo Stato manifesta la sua forza - sia in quella successiva, in cui i patrimoni sottratti ai mafiosi devono essere valorizzati per ritornare alla collettività. Questo intervento, nei suoi due aspetti operativi, deve essere la manifestazione tangibile, in buona sostanza, ancor di più in quelle vaste zone del Sud dove il contrasto alle mafie è lotta di resistenza democratica, della capacità dello Stato repubblicano di essere presente, attraverso quello che ho più volte definito come una sorta di riuso di legalità. Esso deve rappresentare, cioè, una manifestazione dello Stato democratico di esercizio, oltre che del potere di contrasto e controllo, cioè della sua forza, anche e soprattutto, della capacità di mettere a profitto politiche di sviluppo anche mediante il riutilizzo dei proventi di attività criminali. Come ormai la storiografia ha chiaramente evidenziato e diciamolo anche in questa Aula - non sempre lo Stato si è comportato da Stato democratico, in quelle terre che ancora non riescono a recuperare la condizione di sottosviluppo in cui una certa politica di

A dirla in parole semplici, lo Stato, sottratte le risorse (sia essi beni mobili, immobili o aziende) alle mafie, deve poi essere in grado di ridare quelle risorse predate *in primis* alle genti del Sud, per non far minimamente rimpiangere la scelta di stare dalla parte dello Stato democratico repubblicano. Io credo - anche come Italia dei Valori che sull'argomento aveva presentato un disegno di legge di iniziativa popolare, con cui chiedeva che i beni confiscati alle mafie divenissero appunto utili strumenti per raggiungere il bene comune con più penetranti meccanismi per la loro alienazione, se non altrimenti destinati a fini sociali - che l'equilibrio trovato nelle norme che ci apprestiamo ad approvare, per la maggioranza di Governo data, sia il meglio che ad oggi si potesse ottenere. Il provvedimento all'esame, infatti, rappresenta un apprezzabile passo in avanti in grado di correggere i limiti e le inadeguatezze della legislazione vigente (evitando, peraltro che si ripetano nefandezze come quella che ha visto come protagonista il giudice Saguto), con uno sguardo anche di prospettiva attraverso, per esempio, l'estensione delle categorie dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche agli indiziati dei delitti di corruzione nella pubblica amministrazione. Non me ne vogliano quei colleghi che ho appena sentito avanzare sul sul punto alcune critiche, ma ritengo che questa non sia una forzatura, ove non si dimentichi come la storia del contrasto alle mafie ha dimostrato il suo marchio di differenziazione rispetto ad ogni altra associazione criminale è, sì, la sua capacità di relazionarsi con certa classe dirigente, fino a inquinare la politica, ma è anche la facilità con cui riesce a penetrare e condizionare le pubbliche amministrazioni,

Il messaggio lanciato con queste modifiche, si spera, è che il delinquere non paga, perché si finisce in carcere né si consente di accumulare o celare i proventi. Unico rammarico che devo però evidenziare è aver perso, per l'ennesima volta, l'occasione, nel momento in cui si sono modificate le misure personali di prevenzione, di impedire ai sorvegliati speciali per mafia di fare campagna elettorale, per come codificata nel testo di legge che sin dall'inizio di questa Legislatura sto cercando di far approvare, la cosiddetta legge Lazzati, e che si trova impantanata in Commissione affari costituzionali. Ho presentato alcuni emendamenti e un ordine del giorno che spero vengano accolti,

Condivido in pieno, dal punto di vista della tecnica legislativa, la critica rivolta all'aver voluto estendere questi potenti strumenti di contrasto ai cosiddetti reati persecutori e a quelli di terrorismo. Io spero che, con questo, non si indebolisca la funzione primaria

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere la riforma al testo unico antimafia, un provvedimento molto importante per tutto il Paese e soprattutto per la terra dalla quale provengo, la Sicilia. Voglio anch'io, come il relatore, senatore Pagliari, iniziare il mio intervento con il ricordo ed un pensiero alle tante, troppe vittime delle mafie ed un ringraziamento ai cittadini, agli amministratori pubblici, alle associazioni come Libera e a tutti coloro che quotidianamente contrastano la criminalità organizzata. Il provvedimento di cui stiamo discutendo, già approvato alla Camera e modificato in Commissione giustizia, introduce diverse modifiche al codice antimafia, tra le quali quelle relative alla disciplina delle misure di prevenzione personali, alla sorveglianza speciale, all'obbligo di soggiorno e alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali. interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e sulle disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Su questo ultimo punto sono già intervenuta in quest'Aula nel 2014, nel corso della discussione generale sulla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ed è ed è ancora su questo punto che oggi focalizzerò il mio intervento. Nell'intervento in Aula feci delle osservazioni ed anche delle proposte relative sia al mandato che ai criteri di scelta degli amministratori giudiziari e non solo, frutto di esperienze legate alla storia delle aziende sequestrate alla mafia nel mio territorio, esperienze non sempre positive e che in alcuni casi non hanno visto i beni immobili e le aziende confiscate diventare risorse positive ed effettive per la collettività, o in termini di destinazione utile dei beni o in termini di poli produttivi produttivi e forieri di lavoro. Ritengo importante oltre che necessario, oggi più di allora, che le imprese sequestrate siano messe in grado di confrontarsi con il mercato ed abbiano gli strumenti per poter per poter diventare produttive al pari di qualunque altra azienda economica sana, capace di creare lavoro e sviluppo. Il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi con le modifiche apportate dalla Commissione giustizia va in tal senso ed in particolare ed in particolare il Capo III del provvedimento, anche recependo mie valutazioni, modifica proprio la disciplina in tema di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati. Questa parte del provvedimento, infatti, interviene sulle norme che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e sulle norme che regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico, prevedendo che il tribunale, qualora la gestione del bene sequestrato risulti molto complessa, possa nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se essi debbano operare congiuntamente o disgiuntamente. Le modifiche apportate in Commissione, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, recano anche puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Viene riconosciuta inoltre all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuzione. Nel provvedimento in esame vengono altresì introdotti gli strumenti finanziari di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non inquinate dai capitali o dai metodi illeciti. Di grande importanza è l'istituzione presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a partecipare un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, i rappresentanti delle istituzioni (Regione e Ministero dello sviluppo economico) e le associazioni datoriali

agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Viste le modiche che il provvedimento in discussione apporta all'Agenzia nazionale e al suo funzionamento, mi fa piacere ricordare che, accanto ad esempi negativi di aziende rivelatesi prestanome nelle operazioni che l'Agenzia stava effettuando per far riacquisire l'azienda e rimetterla sul mercato, ci sono anche casi virtuosi di riutilizzo. Un esempio davvero importante è costituito da un'azienda della mia provincia (Trapani), la Calcestruzzi Ericina Libera. Vorrei anche rappresentare nuovamente un altro caso di specie, che afferisce ad un'azienda sempre della mia provincia (Trapani), di cui ho conoscenza diretta e per la quale sono intervenuta diverse volte in quest'Aula. Si tratta del Gruppo 6 GDO Srl, con sede in Castelvetrano, azienda in amministrazione giudiziaria dal 2008, che operava nell'ambito della grande distribuzione gestendo direttamente e indirettamente, tramite società collegate e controllate, ovvero avendo concesso a terzi in regime di affitto di un ramo d'azienda, la somministrazione, affiliazione e conduzione di supermercati e *discount* in provincia di Trapani, Agrigento e in parte di Palermo. L'azienda nel 2010 occupava circa 400 addetti, con un fatturato di oltre 120 milioni di euro e con attività in 58 supermercati. A seguito del provvedimento di confisca, tutte le quote societarie sono state trasferite all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Successivamente, il tribunale di Marsala ha dichiarato fallito il gruppo, ritenendo inammissibile l'accordo proposto dall'Agenzia nazionale, che prevedeva la cessione del ramo di azienda, relativo ai punti vendita del Gruppo 6 GDO, ad una società. L'accordo avrebbe consentito la ricollocazione della quasi totalità dei circa 400 lavoratori dei punti vendita direttamente e indirettamente collegati all'azienda castelvetranese della grande distribuzione, con l'avvio immediato dell'attività. Nel novembre 2014 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati ha emanato un decreto che prevedeva, tra l'altro, la riapertura a Castelvetrano dell'ipermercato interno al centro commerciale, con il riassorbimento di una parte dei lavoratori impiegati nel gruppo. Successivamente, quasi tutti i lavoratori della rete della vendita sono stati ricollocati, mentre ad oggi circa 50 lavoratori del centro di distribuzione sono stati posti in mobilità; questa per alcuni è scaduta nel mese di giugno del 2016 e ad oggi risultano purtroppo ancora disoccupati. Signora Presidente, colleghi, concludo con l'auspicio che, con le modifiche che verranno apportate oggi attraverso l'approvazione di questo provvedimento, si riesca ad accelerare quel processo di riforma dell'istituto dell'Agenzia, divenuto ormai indispensabile, affinché casi come quello del Gruppo 6 GDO e non solo non si ripetano, e che il prezzo della crisi economica, che ha generato disperazione e perdita di lavoro ovunque, non sia pagato doppiamente da quei lavoratori onesti - e voglio sottolinearlo: onesti - che, prestando la loro opera in un'azienda confiscata alla mafia, vedono i loro diritti doppiamente messi in pericolo. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché non si consolidi il messaggio secondo cui la mafia dà il lavoro e lo Stato lo toglie. Per questo dobbiamo adoperarci per far sì che le aziende confiscate continuino ad offrire lavoro e a produrre e che i beni confiscati diventino di utilità sociale, direttamente o tramite l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla loro smobilitazione; in tal senso, il codice fa un notevole passo in avanti.

dal versante delle interdittive antimafia, che sono atti amministrativi, mi sono guadagnato sul campo un avviso di garanzia con l'aggravante mafiosa; e questo non perché io conosca qualcuno della mafia o della 'ndrangheta, direttamente o indirettamente, ma perché qualcuno ha semplicemente opinato che le opinioni espresse in Aula, in Commissione o in Commissione antimafia, ripetute all'esterno, in una dialettica con le prefetture e con chi, secondo me in maniera sbagliata, interpretava queste norme, diventano automaticamente qualcosa da qualcosa da marchiare con l'aggravante, anche se i rapporti sono stati con Gratteri, con Cantone, con i prefetti, con la polizia e con i carabinieri, quindi solo nel circuito della legalità. A quanto pare in Italia basta

ciò che il Parlamento sta facendo, se si comporta in questa maniera - dove si dice che stiamo lavorando per affinare i meccanismi di contrasto alla mafia per far sì che i sequestri dei beni mafiosi vengano gestiti con intelligenza e non si ripetano i casi Saguto, a cui abbiamo assistito a Palermo. Mi

modifica l'articolo 4 del codice antimafia inserendo nuovi soggetti tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno e l'obbligo di soggiorno.

stiamo votando provvedimenti che cominceranno con il sequestro di tutti i beni a carico del malcapitato assessore, sindaco o amministratore pubblico, e poi passeranno trent'anni trent'anni nei quali i magistrati riterranno se proclamarlo innocente o colpevole. Intanto faccio presente che il sequestro dei beni è un fatto gravissimo,

allargare eccezionali misure contro la criminalità organizzata a migliaia e migliaia di pubblici amministratori. Vorrei sapere quale kamikaze domani si metterà a fare il sindaco o l'assessore sapendo di avere sulla testa una spada di Damocle.

Abbiamo inserito, o meglio hanno inserito - io ero contrario - tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione anche gli indiziati del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640*-bis*

misure di prevenzione personali si applicano anche a coloro che compiono atti esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista. Anche questo non ho capito bene cosa c'entri. Colleghi, mi sono avvalso dell'aiuto di tecnici che hanno seguito il testo, perché non è sempre facile capire quello che scriviamo. sono le norme venute oggi all'attenzione del Senato; norme che, appunto, spaziano dai reati contro la pubblica amministrazione al problema del terrorismo, agli atti persecutori, fino ad

E sarei altrettanto lieto di sapere se il Governo e la maggioranza, anche alla luce dei risultati elettorali dell'altro giorno, vogliono continuare a sfornare leggi - l'ultima, per esempio, è la riforma del codice penale - che hanno raccolto la totale

stante un collegamento con attività mafiosa, che però non c'è. Là dicevano che c'era ed era sicuro che ci fosse; qui invece abbiamo dimostrato che non c'è. Ci sarà?

alla luce di come sono stati accolti altri provvedimenti, ci sarebbe leggermente da vergognarsi. Spero, comunque, che ci sarà tutto il tempo per rimediare a questi errori. Signora Presidente, «Emotivo, episodico, fluttuante. Motivato solo dall'impressione suscitata da un dato crimine o dall'effetto che una particolare iniziativa governativa può esercitare sull'opinione pubblica»: così Giovanni Falcone descriveva l'impegno dello Stato nel combattere la mafia. Errori di valutazione, inefficacia delle azioni di contrasto, assenza di volontà politica: tutte cose che hanno segnato numerose fasi della storia dell'antimafia in Italia, garantendo ai *clan* la libertà di agire pressoché indisturbati per anni, libertà di agire che ha permesso di trarre dall'abbattimento dei tempi e delle fatiche il guadagno e il successo tanto nelle carriere personali, quanto nelle realtà aziendali che scelgono di utilizzare i servizi illeciti. La mancanza di incisività e presenza dello Stato, la lentezza e le inefficienze vengono considerate, a tutti gli effetti, concause responsabili dell'esposizione e dell'espansione delle organizzazioni criminali. Si limita il successo di chi rispetta tutte le regole se non si contrasta chi sistematicamente le infrange; una lentezza che, nel migliore dei casi, porta a una tolleranza subdola e che ha portato a tenere nel cassetto l'approvazione di una legge sui reati ambientali, mentre le cosche mafiose imperavano nella terra dei fuochi. E' proprio nel contrastare questo imperversare che, negli ultimi anni, abbiamo registrato fasi di successo dello Stato e fasi in cui la criminalità organizzata ha preso una grande forza; forza derivata da due fattori: la capacità di adattamento e una marcata resilienza, che riconosciamo ai metalli di assorbire un urto senza rompersi. Nuove fonti di arricchimento hanno guidato le cosche mafiose in territori profondamente differenti, servendosi di reti clientelari, corruttive e criminali preesistenti. In una società sempre più liquida, dove le comunità si trovano in crisi e le organizzazioni sono prive di parte del loro potere, le moderne mafie si stanno rivelando una realtà estremamente solida e duratura. È la capacità di adattamento di queste realtà che ci spinge ad affrontare il problema mafioso; è la presenza di un nemico così abile che non ci permette di interpretare ciò che accade, di ripetere gli errori commessi in passato e di agire tardi. «Non credo che lo Stato italiano abbia veramente l'intenzione di combattere la mafia»: se questa affermazione del pentito Tommaso Buscetta corrispondesse al vero, oggi non saremmo certo qui a discutere di questo

modifica alla disciplina delle misure di prevenzione personale, dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione, rende più efficaci e tempestivi l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale, patrimoniale, il sequestro e la possibilità del controllo giudiziario delle aziende. Vi è poi maggiore attenzione e trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro; modifica il regime della tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali; riorganizza l'Agenzia nazionale dei beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Introduce misure in contrasto al caporalato: è importante per le aziende sequestrate e confiscate favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali. Ed è proprio questa, signora Presidente, la chiave del successo. Con l'aiuto di provvedimenti di questo tipo bisogna sfidare le mafie proprio laddove operano; sfidarle sul terreno dell'economia, del sociale, sulle attività dove costruiscono alternativa alla legalità. sfidare le mafie dove trovano consenso con la bonifica delle aziende e dell'economia locale. Le confische e il mantenimento della forza lavoro ottengono un duplice risultato: dimostrare che si può sconfiggere la mafia con azioni che trasformano i beni strumento dell'azienda criminale in nuove opportunità di legalità, nella sensazione di libertà

Emersione della legalità e affossamento dell'azione criminale non possono, però, rimanere, signora Presidente, sulla carta. controlli, prevenzione e azioni repressive. La mafia dà la sensazione, molte volte, troppo spesso, di poter gestire tutto a piacimento e con una semplicità disarmante. La mafia continua a essere

le mani sui supermercati e su società di vigilanza; arresti tra Catania e Milano; arresti per mafia per il *business* dei migranti di Isola di Capo Rizzuto; arresti per mafia nel settore delle estorsioni a Termini Imerese; arresti per mafia a Catania per droga e sequestro di società nel settore della raccolta dei rifiuti e nei bar, ristoranti e negozi di abbigliamento per svariati milioni di euro; arresti per mafia a Messina per traffico di stupefacenti, estorsioni, furti e rapine. Presidente, il provvedimento è diretto a modificare la disciplina prevista al fine di rendere ancora più efficace ed efficiente la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e per rendere più celere la loro destinazione dopo la confisca.

aziende con le quali le associazioni criminali si arricchiscono e finanziano l'organizzazione e la loro attività. Se noi, signora Presidente, con un provvedimento di questo tipo e con l'aiuto della magistratura e delle Forze dell'ordine, che io ringrazio nuovamente,

Signora Presidente, onorevoli senatori, è passato troppo tempo - quasi due anni, dall'11 novembre 2015 - da quando il disegno di legge che oggi giunge qui nell'Aula del Senato ha ricevuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento; un tempo eccessivo, smisurato che - come accade spesso nella vita parlamentare - ha accresciuto nell'opinione pubblica più attenta ed esigente il sospetto e la preoccupazione che anche questa volta il legislatore non ce l'avrebbe fatta, facendo nuovamente marcia indietro, rinviando *sine die* un provvedimento così utile al nostro Paese. E addirittura, nella propaganda che di tanto in tanto gonfia la voglia irresponsabile di andare al voto anticipato costi quel che costi - si è corso il rischio di dimenticarsi dell'importanza assoluta di portare a rapido compimento il progetto di riforma del sistema della giustizia. Così, il lavoro della Commissione giustizia - desidero ringraziarla per aver proceduto a un esame minuzioso del testo trasmesso dalla Camera - è stato spesso intralciato da insidie esterne, da continui rinvii, da *stop and go* e da un clima nervoso tanto che solo all'ultimo, con uno scatto finale, è stato possibile concludere positivamente l'esame sul testo. Nel frattempo abbiamo ricevuto le giuste sollecitazioni a fare presto e bene da ARCI, Libera, CGIL, ACLI, Avviso Pubblico e da altre associazioni che hanno elaborato la proposta

che meno di quindici giorni fa ci ha giustamente messo in guardia da eventuali passi falsi, sostenendo chiaramente che senza il nuovo codice ci si arrende alla corruzione.

l'associazione Transparency International ci ha assegnato uno dei peggiori risultati tra le democrazie europee, posizionandoci centoventesimi su 138 Paesi per quanto riguarda i favoritismi nelle decisioni dei dipendenti pubblici per quanto riguarda la distrazione di fondi pubblici. Eppure, in questa legislatura il Parlamento ha fatto passi avanti importanti nella lotta contro la corruzione e le mafie, approvando le nuove norme sullo scambio elettorale politico-mafioso, sul falso in bilancio, sui reati ambientali, sul caporalato, sul nuovo codice dei contratti e degli appalti, nonché, da ultimo, sulla riforma del codice penale e di procedura penale. Oggi il Senato può votare un testo equilibrato e di prospettiva, che migliora ulteriormente il lungo lavoro svolto dalla Camera e offre una sintesi positiva per correggere i limiti e le inadeguatezze del vecchio codice antimafia, il decreto legislativo n.159 del 2011, del resto già definito giustamente un'occasione perduta. Il provvedimento che oggi discutiamo intende, quindi, assumere volutamente una portata risolutiva. Si presenta come un testo molto complesso, in cui si modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; si interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni

e 316 del codice penale. In questo modo sequestri e misure contro i beni della mafia potranno essere applicati anche ai corrotti. Tra le norme più importanti desidero ricordare le nuove disposizioni che intervengono sulle norme del codice antimafia per definire i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. L'esame in Commissione giustizia non ha apportato alcuna particolare modifica di rilievo rispetto alla disposizione in oggetto presente nel testo già approvato dalla Camera dei deputati. Su quest'aspetto è stato compiuto un lavoro di sintesi, anche se avrei auspicato che i criteri di nomina degli amministratori giudiziari non venissero delegati ad alcun decreto successivo del Governo, ma potessero essere precisati già nel testo del disegno di legge, o che l'iscrizione all'albo fosse subordinata anche al possesso del requisito di onorabilità oltre che ai criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza, per valutare correttamente i diversi profili dei professionisti da incaricare. Una valutazione positiva può essere compiuta anche per le nuove norme che disegnano la nuova struttura dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati. L'obiettivo è colmare un ritardo normativo che risale alla legge in materia del 1996, mentre il varo dell'Agenzia è arrivato solo quattordici anni dopo, nel 2010. Oggi occorre cominciare a ripensare la filosofia di fondo, considerando i beni sottratti alle mafie come risorse. Per questo non sono più tollerabili sprechi di denaro pubblico o tempi biblici come purtroppo viene svelato costantemente da diverse inchieste - affinché i cittadini siano messi nella condizione di percepire concretamente che la legalità conviene. Il nuovo codice inserisce, inoltre, positivamente anche la nuova confisca allargata, estendendo - da un lato - il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere e - dall'altro - escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato

a seguito dell'omicidio di Giovanni Falcone (23 maggio 1992) che veniva emanato il decreto. Poi, nell'*iter* di conversione, veniva compiuto l'omicidio di Paolo Borsellino (19 luglio 1992). La *ratio* della norma, che viene mantenuta ed estesa, sta tutta in questa nobile pagina dell'antimafia. Nel testo in esame, infatti, si prevede la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Così, tra i nuovi delitti per cui si può procedere alla confisca allargata, figurano il disastro ambientale, l'associazione finalizzata alla commissione di reati ambientali, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, l'autoriciclaggio e il traffico illecito di rifiuti.

laddove sono indicati i soggetti che devono dotarsi, richiedendola alle prefetture competenti per territorio, della documentazione antimafia, costituita dalla comunicazione e dall'informazione (in una parola: i certificati). Ebbene, nel caso di imprese consorziate, attualmente si prevede che l'obbligo di richiedere i certificati grava, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, sul legale rappresentante e sugli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché su ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore

non stimolano nelle prefetture alcun tipo di verifica su presenza o condizionamento mafioso nella compagine sociale o consortile. Franco Roberti ha chiaramente affermato che si tratta di una grave lacuna perché, attraverso le forme consortili, le imprese espressione delle cosche mafiose possono agevolmente eludere il sistema dei controlli, pur altrimenti molto sofisticato. Oggi, anche con il voto di quest'emendamento in Aula, possiamo migliorare ulteriormente il disegno di legge, raggiungendo un risultato molto significativo. Credo ne valga la pena, perché l'Italia e i più giovani meritano un futuro di libertà e di riscatto dalle mafie. Signora Presidente, ci troviamo davanti a un provvedimento estremamente tecnico, un provvedimento necessario che ha avuto un lungo *iter*

Non so fino a che punto sia più efficace il discorso tecnico o quello culturale. Quello che so per certo è che gli aspetti culturali della lotta contro la mafia non si

contro la mafia, sono i più importanti interpreti della lotta culturale contro l'illegalità e, di conseguenza, contro quel terreno fecondo in cui radica la criminalità organizzata. Penso

E penso che la diseguaglianza non sia sufficientemente combattuta da questo Paese. Penso che la mafia si rafforzi nel caos amministrativo,

purtroppo riguardi tutti gli aspetti della quotidianità delle persone che in questa condizione non possono che vedere nello Stato un qualcosa di estraneo, lontano, ingiusto e inefficace.

Penso che la propagandata flessibilità, che oggi è diventata in realtà precarietà, sia un grande regalo alla criminalità organizzata proprio nella mancanza di certezza di quello che si è, delle proprie entrate, delle risorse future per mantenere sé stessi e la propria famiglia, la criminalità organizzata, che in realtà è estremamente ben organizzata, si rafforza.

Ma credo altresì molto difficile che sia appetibile l'opzione della legalità quando ci sono delle differenze così grandi e quando chi vive nella giustizia e nella legalità si ritrova a dover vivere in condizioni di difficoltà. Ho recentemente visitato il carcere di Parma, che è nuovamente

in cui i famigliari dei detenuti non vadano a colloquio; ci sono dei detenuti molto anziani, anche ultranovantenni, la cui famiglia non ha mai mancato un incontro. E noi sappiamo che essi

Lo dice anche Gratteri: la 'ndrangheta si nutre di simboli, di simboli forti. Nel carcere di Parma, sulla carta, ci sono 400 unità della polizia penitenziaria. In realtà, gli effettivi sono 250 e si arriva, per tutta una serie di meccanismi, a una riduzione dell'organico tale per cui, di notte, la sicurezza del carcere di Parma è garantita da sole undici unità della polizia penitenziaria.

come un insegnante: credo siano entrambi ruoli importanti e anche fortemente simbolici. Non sto dicendo che lo Stato debba competere

dai più giovani. Credo sia una responsabilità profonda quella di chi oggi deve fare in modo che lo Stato funzioni bene.

Purtroppo la cronaca ci rimanda comunque a una fetta dello Stato che non è al di sopra dei sospetti.

Se ciò non viene profondamente percepito nella cultura del *civil servant*, in tutti i luoghi in cui lo Stato manifesta se stesso, dal più modesto al più alto, allora la lotta contro la mafia non è neanche cominciata.

l'approvazione del nuovo codice antimafia è ormai in dirittura d'arrivo. È stato indubbiamente un *iter* complesso, che ha impegnato la Commissione giustizia quanto la Commissione antimafia per quasi quattro anni. Nonostante ciò, permangono alcune riserve in merito all'efficacia delle disposizioni che andranno a novellare il codice descritto dal decreto legislativo n. 159 Il codice del 2011, infatti, ha mostrato da subito, al di là delle buone intenzioni che hanno animato la sua entrata in vigore, diverse criticità. Ne sono esempio la complessità del testo e un eccesso di burocrazia, che hanno vanificato l'intento che lo Stato si era prefisso di realizzare: dotarsi di una efficace normativa in materia di sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose e del riutilizzo sociale degli stessi. È quindi lecito, dopo questa esperienza, domandarsi se l'obiettivo che ci siamo prefissi di raggiungere con questa revisione del codice antimafia potrà essere concretamente realizzato. La creazione dei due fondi di garanzia (uno in favore delle imprese e l'altro per la crescita sostenibile), l'allargamento della platea dei destinatari delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, l'inserimento di un importante distinguo tra l'istituto del controllo giudiziario (che non prevede l'ablazione dei beni) da quello dell'amministrazione giudiziaria sono interventi che vanno nella giusta direzione. Anche l'annoso problema degli amministratori giudiziari è stato messo in discussione, soprattutto per ciò che riguarda i compensi eccessivamente onerosi e il cumulo di incarichi, condizioni che hanno gettato troppe ombre sull'operato dello Stato nella lotta alla mafia. Già da questa breve disamina si può desumere che le disposizioni del disegno di legge n. 2134 rappresentano un drastico ripensamento del lavoro svolto nel 2011. Malgrado ciò, il provvedimento poteva essere maggiormente incisivo, non tanto per quanto concerne le singole disposizioni ma nella sua prospettiva d'insieme. È l'esperienza pregressa, infatti, a suggerirci che non è la somma dei singoli interventi ad indicarci la loro efficacia, quanto l'organicità degli stessi. Nella lotta alla criminalità organizzata lo Stato si muove purtroppo su un terreno impervio, reso ancora più difficoltoso dal fatto che la mafia è radicata sul territorio nazionale da moltissimo tempo mentre, per diverse ragioni, le istituzioni fino ad ora si sono mosse con molto ritardo e con un fare incerto. Quando parliamo di mafia, infatti, ci riferiamo ad un'economia sommersa che secondo stime confermate dal Governo, incide sul PIL per il 12,4 cento, con circa 60 miliardi di euro di risorse che ogni anno vengono sottratte allo sviluppo e alla crescita economica nazionale. L'obiettivo da raggiungere è di togliere alla mafia le risorse economiche che la mantengono in vita. Se aggrediamo cosa nostra sul piano economico le togliamo la sua stessa ragione d'esistere, dal momento che il fine della criminalità organizzata è quello di arricchirsi attraverso il controllo di realtà industriali e commerciali dedite al riciclo di denaro sporco. In questo conflitto lo Stato può avere la meglio solo allargando le maglie della legalità, per creare sviluppo e crescita economica. Ecco perché una nuova e più incisiva normativa per amministrare i beni confiscati alla criminalità si è resa necessaria per non ripetere gli errori di un recente passato, ovvero privare di valore le confische. In questo modo è stato creato un danno allo Stato, ma anche a quei patrimoni che, in caso di proscioglimento o assoluzione, sarebbero ritornati al legittimo proprietario. Ciò che accaduto fino a questo momento è stato l'esatto contrario. Non basta togliere alla mafia; è necessario che quei beni diventino una rendita attraverso cui è possibile avere maggiori risorse per il contrasto della criminalità. Senza adeguati accorgimenti, infatti, lo Stato finirà per soccombere nella lotta all'economia illegale, a cominciare dalla questione lavoro. Sono migliaia le persone che, a loro insaputa, lavorano alle dipendenze della mafia. Quando lo Stato interviene con la confisca delle aziende, il lavoro dei dipendenti diventa a rischio, anzitutto perché la notizia stessa del sequestro crea nell'immediato panico e sconcerto, nei dipendenti ma anche tra i fornitori e i creditori. È questa perdita di fiducia a provocare automaticamente la crisi aziendale, che pregiudica la sopravvivenza dell'attività. Ed è a questo punto che l'amministrazione giudiziaria dovrebbe intervenire in maniera intelligente. Se il sequestro non è definitivo è necessario essere lungimiranti e non far perdere di valore l'attività. Nel caso di confisca definitiva, invece, la scelta deve essere o di vendere l'azienda oppure di agire in regime di continuità, senza creare crisi interne e generare licenziamenti. Va riconosciuto a questo testo il merito di aver introdotto nuovi strumenti per il rilancio delle imprese sequestrate o confiscate, ad esempio per garantire linee di credito interrotte, sgravi fiscali e un accesso agevolato agli ammortizzatori sociali. Rimane tuttavia un dubbio, quello sulla realizzazione di queste previsioni di legge. Anche se sono stati definiti i tempi per i procedimenti, è alquanto probabile che senza maggiori risorse umane queste tempistiche rimangano tali soltanto sulla carta. Il fattore umano nella lotta alla criminalità organizzata è imprescindibile, poiché solo professionalità esperte e con una profonda conoscenza delle problematiche territoriali possono prendere le scelte più appropriate, trattando casi simili con soluzioni diverse sulla base della realtà in cui i beni incidono. La lotta alla mafia non è soltanto far emergere la legalità: in gioco c'è la credibilità stessa dello Stato. Dove lo Stato lascia territori senza un valido contesto economico e occupazionale la mafia riesce ad insidiarsi, tanto che in molte zone del Paese c'è chi pensa che la mafia crei più posti di lavoro dello Stato, quindi che sia più affidabile delle promesse delle istituzioni. In tal senso, purtroppo, il Sud è maggiormente esposto nei confronti del resto del Paese. Nel Meridione, con una disoccupazione che raggiunge picchi di oltre il 60 per cento, le attività criminali rischiano di essere considerate dai cittadini un'alternativa allo Stato che crea occupazione. Troppo spesso è capitato che quando lo Stato è intervenuto nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata si sia determinata la crisi di aziende che erano ancora in grado di produrre, togliendo al territorio ricchezza ed occupazione. Questo è il vero fallimento cui andiamo incontro se non sostituiamo alla produttività generata dalla criminalità un'economia legale sostenuta dallo Stato. Nel frattempo i cittadini, a ragione, si sentono abbandonati dalle istituzioni che avrebbero dovuto difenderli. In questo senso, il sequestro dei beni è l'inizio e non la fine di un procedimento molto complesso teso a salvaguardare le comunità locali.

«si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni». Signora Presidente, mi rivolgo essenzialmente ai relatori e al Governo,

legislatura per l'approvazione del decreto legislativo n. 159 del 2011, ossia il codice antimafia che abbiamo fatto dopo aver stabilizzato penitenziario e aver dato una disciplina che, con l'articolo 2 del disegno di legge sulla sicurezza, ottenne l'unanimità del Parlamento. Ci sono alcune modifiche che possono essere utili, ma, quando la modifica che viene apportata peggiora il testo, allora bisogna stare molto attenti. Noi abbiamo una prima questione: attenzione a non diminuire il valore del codice antimafia. La mafia necessita di una disciplina particolare, se vogliamo combatterla veramente, una disciplina giudiziaria e giuridica di tutti gli interventi che rispondono all'esigenza di estirpare un cancro nel nostro Paese e che si applica alle associazioni organizzate di tipo mafioso. Quando però si allarga il campo di applicazione, si rischia di incorrere in violazioni dei principi di civiltà giuridica.

probabilmente non si è riflettuto molto sulla questione. Perché? Noi innanzitutto dobbiamo tener conto del fatto che per tutti i reati indicati nell'articolo 4 del codice antimafia deve sussistere la pericolosità sociale. Cito soltanto l'ultima delle sentenze della Corte di cassazione, la sentenza n. 50128 del 25 novembre 2016: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità

che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione». Ne ho citata una, ma i principi giuridici che sono alla base di questa decisione sono conformi in tutte le decisioni della Corte.

sociale. Non stiamo parlando di un appartenente all'associazione mafiosa, per cui anche la Corte di cassazione ha detto che, ancorché si tratti di concorso esterno o ancorché si tratti di un semplice partecipe all'associazione, per questi motivi c'è la sussistenza della pericolosità sociale, a meno che non risulti una rottura con quello che era il suo passato rispetto ad oggi. Qui noi non ci troviamo di fronte a una

di aver commesso un reato. Si può applicare il codice antimafia? Si può dire che il tizio, che è indiziato di aver commesso forse anche un reato

né di accertamento di responsabilità, né di indagine. Per cui arriviamo in ipotesi ad applicare misure personali o addirittura la confisca nei confronti di soggetti non condannati.

E come facciamo a coniugare un'ipotesi di valenza dell'indiziato rispetto a un'ipotesi di successiva assoluzione, sempre che fosse successivamente indagato? Il testo, infatti, non lo dice:

è possibile fare una correzione? Non ho presentato emendamenti. Do l'indicazione di un problema serio. Non cito i vari giuristi intervenuti in questo fine settimana su questa materia e che tutti avete letto, ma tutti hanno messo in evidenza i problemi che sorgono da un punto di vista giuridico-costituzionale. Credo che un minimo di riflessione dobbiamo farla tutti. Vengo alla seconda questione. Voi

Trapani? Queste due eccezioni sono inspiegabili. Probabilmente sarebbe corretto eliminarle, tanto la regola generale del capoluogo del distretto avrebbe la sua valenza.

le funzioni di competenza spettanti al procuratore della Repubblica sono attribuite al procuratore della Repubblica. Questo avevamo scritto. Oggi mi dite «anche» al procuratore della Repubblica, previo coordinamento. In tal modo andate ad alterare quel rapporto, che avevamo costruito insieme, di funzionalità perché significava evitare problemi di accavallamento di competenze.

La competenza del procuratore del circondario dove dimora la persona proposta e la competenza del procuratore del distretto - e lì anche del procuratore della Repubblica - per quanto concerne la mafia: questa era la logica del provvedimento. Non ho capito perché andiamo ad alterare un sistema che è stato frutto dell'elaborazione comune e che ha dato buoni risultati.

le coperture di bilancio e quindi siete stati costretti a escludere il concorso e a limitarvi soltanto alla mobilità. Siccome già sei sedi diventavano una cosa non coerente perché non funzionano, che cosa avete fatto? Avete ridotto il tutto non più al concorso per la metà, ma la scelta di professionalità eccezionali avviene attraverso la mobilità.

deve essere composta da persone in gamba perché abbiamo 17.000 immobili confiscati e che non vengono gestiti secondo quelle che sono le regole!

è l'affermazione del principio di legalità anche nella gestione dei beni confiscati. Dobbiamo partire da un presupposto: nel nostro sistema non ci sarebbe corruzione, signor Sottosegretario, se si riducessero l'ambito e l'area di discrezionalità amministrativa.

i controlli e la loro funzionalità. I controlli servono a evitare la corruzione e i reati che si basano sulla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Eppure, dal punto di vista giudiziario - lo ha ricordato il ministro Orlando in quest'Aula - sono pochissime, anzi quasi nulle in molti tribunali,

abbiamo commemorato Stefano Rodotà. Era una delle cose che diceva quando si discuteva di corruzione,

trasparente e coerente con i compiti che la legge e la Costituzione le assegna, evitando che qualcuno possa approfittarne. Signora Presidente, cari colleghi, la confisca dei beni ai mafiosi è un fondamentale strumento di lotta alla criminalità organizzata, perché vanifica l'accumulazione illecita di beni e capitali e, di conseguenza, mette in ginocchio le economie non solo di alcune Regioni d'Italia, ma di tutto il nostro Paese, ledendo oltretutto l'immagine e la credibilità di una società intera. In mancanza di finanza mafiosa - chiamiamola così - e sgominata l'economia della criminalità, ci avvicineremo all'obiettivo di sradicare le maledette mafie, che sono evidentemente le principali responsabili di alcune delle più grandi carneficine e di una delle più profonde depressioni economiche. Ormai siamo già decisamente avanti nella lotta sempiterna al crimine organizzato. Il grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle Forze dell'ordine stanno conseguendo successi sempre maggiori su questo terreno, tanto che l'entità del patrimonio confiscato sembra aver raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro e cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevanti, che sempre più frequentemente si succedono. Tale fatto comincia a impegnare fortemente le strutture dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e rende la loro gestione sempre più onerosa e complessa per lo Stato.

Finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali, ma la situazione che si sta venendo a creare pone diversi problemi. alla necessità del rafforzamento dell'Agenzia, fondamentale strumento per l'amministrazione di tale compendio, nonché all'accelerazione dei tempi per la consegna a enti locali e associazioni (quelli che ne facciano richiesta in tempi rapidi) dei beni congeniali alle loro attività. La messa a frutto attraverso la vendita a stima di mercato e certificata dalle strutture pubbliche dei beni mobili e di quelli immobili non richiesti o non congeniali; un regime agile e certo di gestione delle aziende interessate in quanto sottratte ai mafiosi per restituirle ad una economia sana, quella che garantisce il benessere dei nostri concittadini. Però, a parte queste esigenze gestionali e contabili, c'è da rilevare che lo Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l'insieme degli interessi pubblici della collettività. È necessario dunque reperire sempre maggiori risorse malate per arrivare ad un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al contempo per affrontare un'emergenza finanziaria senza precedenti cui la criminalità di stampo mafioso non solo - ripetiamo - non è estranea ma di cui spesso è una delle cause prime. Quindi, un migliore e più razionale utilizzo dei beni confiscati alla mafia e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe, *in primis*, di non abbassare la guardia nel contrasto dell'illegalità e di perseguire obiettivi pubblici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico per scongiurare lo sforamento del rapporto *deficit*-PIL, pagare finalmente i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, che - come vediamo anche in questi giorni - è tema di grandissima attualità,

avvelenati dalle ecomafie e per mettere in sicurezza i territori a rischio idrogeologico, dunque, sarebbe per la criminalità uno smacco mortale. L'obiettivo resta, dunque, quello di migliorare il codice antimafia orientando la destinazione delle risorse, per restituire finalmente al Paese i beni illecitamente raccolti dai mafiosi, riportandoli nella disponibilità del cittadino onesto, spesso vittima designata dell'odioso furto di futuro da parte dell'antistato.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, a distanza di sei anni dalla sua introduzione, era giunto per il nostro Paese il momento di una revisione del codice antimafia, una legge concepita con alte ambizioni che, ben presto, si è rivelata limitata e parzialmente inadeguata rispetto al fine di migliorare le azioni di contrasto alla criminalità organizzata. Numerosi sono stati negli anni i rilievi pervenuti all'attenzione del Parlamento da parte di magistratura, Forze dell'ordine e addetti ai lavori, sino a spingere il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, a definire il codice una occasione perduta, non essendo riuscito né nell'intento di rafforzare le azioni di contrasto, né nel realizzare l'obiettivo di armonizzare l'intera disciplina in materia di criminalità organizzata, limite che caratterizzava la normativa antimafia precedente. Ora, dopo ulteriori mesi di ritardo, con il testo approvato alla Camera addirittura nel 2015 e arenatosi per troppo tempo in Commissione giustizia qui al Senato, ci troviamo finalmente in Aula con una normativa che è sintesi di un lavoro durato mesi da parte della Commissione parlamentare antimafia, di cui mi onoro di far parte. All'interno della Commissione, dopo aver approvato una relazione sulla riforma del sistema di gestione dei dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, abbiamo effettuato, grazie agli spunti ricevuti durante numerose audizioni effettuate con cadenza settimanale, una serie di modifiche al codice, al fine di semplificare la disciplina delle misure di prevenzione e di assicurare procedure più snelle e coordinate e adatte alla gestione dei beni confiscati, recependo anche le indicazioni che emergono fatte pervenire dalla magistratura. L'aggressione ai beni della criminalità organizzata e la loro confisca, nei casi previsti dalla legge, rappresenta, infatti, uno strumento essenziale nella lotta alla mafia perché attacca direttamente l'accumulazione illegale di patrimoni. L'entità del patrimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro. Tra i principali compiti di uno Stato, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei propri cittadini, vi è certamente l'obbligo di mettere in piedi un efficiente sistema normativo di contrasto alla ricchezza e di aggressione dei patrimoni illeciti, uno strumento ineludibile nella lotta al crimine organizzato. Combattere l'illegalità economica significa, quindi, prima di tutto aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, restituirli alla collettività e porli alla base della costruzione di nuove relazioni economiche sane e legali, che pongano il lavoro e la dignità delle persone al centro di un nuovo percorso di riscatto civile e sociale. Quando però oggetto del sequestro è un'azienda, nel passaggio dal circuito illecito a quello legale questa rischia di fallire o di chiudere a causa della mancanza di strumenti adeguati a sostegno del difficile percorso di riemersione alla legalità. Ci troviamo pertanto di fronte a un triste paradosso: tante attività economiche per anni nelle mani della mafia, dopo il sequestro, anziché divenire modelli di legalità economica, falliscono. In trentacinque anni di lotta ai patrimoni mafiosi, a partire dall'introduzione della legge Rognoni-La Torre, decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici in tutto il territorio nazionale, in tutti i settori produttivi e in tutte le aree geografiche del nostro Paese, hanno perso il lavoro. Purtroppo, infatti, troppo spesso l'applicazione della misura di prevenzione provoca l'allarme dei clienti (che si rivolgono ad altre aziende), dei fornitori (che tendono a richiedere immediatamente il saldo dei pagamenti dovuti), delle banche (che chiudono i rubinetti del credito). Ciò avviene proprio in territori già fortemente condizionati dalla criminalità organizzata: le Regioni con il numero più alto di aziende sequestrate e confiscate sono infatti quelle del Sud Italia, Sicilia e Campania in testa, ma anche il Lazio e la Lombardia, e poi di nuovo al Sud, con la Calabria. Questa situazione rischia di diventare uno dei simboli della sconfitta dello Stato nei confronti della criminalità, che spesso ha posto alla base del suo consenso la capacità di garantire lavoro e reddito, seppur illegale, in territori flagellati da disoccupazione ed esclusione sociale. Il ritorno alla legalità deve invece rappresentare un volano per lo sviluppo economico e non un ulteriore impedimento alla prosecuzione dell'attività produttiva, soprattutto visto il periodo di grave crisi economica che l'Italia attraversa da anni. Per questo, nello specifico, il provvedimento che oggi discutiamo, già approvato dalla Camera dei deputati e che lì dovrà tornare dopo le tante modifiche espresse dalla Commissione giustizia, è un testo frutto di un lunghissimo lavoro e che riunisce sei proposte di legge di iniziativa parlamentare e una proposta di iniziativa 36 articoli, suddivisi in due macro parti, la prima delle quali ridisegna il meccanismo delle misure di prevenzione e introduce lasciatemelo dire - una radicale, straordinaria novità per il nostro ordinamento: le misure di prevenzione, soprattutto patrimoniale, già previste contro i beni della mafia saranno finalmente applicate anche a chi si macchia di reati contro la pubblica amministrazione. Sono inoltre ben felice di ricordare che rispetto al testo uscito dalla Camera, in Commissione l'ambito soggettivo di applicazione è stato esteso anche ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e ai delitti di atti persecutori, tra cui lo *stalking* che, come ha giustamente ricordato il senatore Lumia durante la sua relazione, è uno dei reati che meglio si combatte con attività di prevenzione. Se attraverso questa modifica potremo aver salvato anche solo una possibile vittima di femminicidio, quello conseguito oggi in quest'Aula sarà, già solo per questo, un risultato storico. La seconda parte della riforma, invece, modifica la disciplina attuale della gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e la successiva destinazione a seguito della confisca, introducendo significative modifiche

a criteri di efficienza ed economicità. Il testo, quindi, si occupa sia dell'applicazione delle misure di prevenzione sia della gestione della destinazione dei beni confiscati. Due situazioni distinte e successive, ma strettamente collegate tra loro. Lo scopo del testo, dunque, è quello di garantire l'efficacia delle misure di prevenzione nell'ambito dell'azione di contrasto alle attività mafiose, tutelando al contempo i lavoratori coinvolti e assicurando una *governance* dell'azienda tesa alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Le modifiche al Libro I del codice antimafia, dedicato alle misure di prevenzione, dovranno nel complesso rendere più efficace

si parte dal reato all'apparenza meno grave, se paragonato a omicidi, *racket*, o traffico di droga, ma che mina dalle fondamenta il buon andamento di una società. Ottima, inoltre, l'istituzione di sezioni o di collegi specializzati, chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice antimafia. Dobbiamo, infatti, fare di tutto per favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, dobbiamo prevedere misure incisive, come l'istituzione di un fondo e altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali, magari attraverso la previsione di sgravi per chi assume *ex* dipendenti di aziende sottoposte a sequestro o a confisca rimasti senza lavoro. Infine, si è ritenuto necessario riorganizzare e potenziare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, che rimane sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e della quale sono state istituite nuove sedi periferiche; oltre Reggio Calabria anche Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano. Al fine di combattere episodi di corruzione e malversazione di denaro pubblico, e a seguito degli scandali verificatisi in Sicilia, si è poi deciso di garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, assicurando competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e rotazione degli stessi. Colpire i patrimoni della criminalità organizzata non è però sufficiente se a quest'azione non si accompagna la restituzione degli stessi beni alla collettività e il loro utilizzo per scopi produttivi. La perdita di posti di lavoro e la conseguente instaurazione di un clima di tensione sociale non consentono un contrasto

lo Stato non riesce nello stesso obiettivo. Sulla base di queste considerazioni mi auguro che in futuro si possano studiare nuove e più efficaci proposte per il riutilizzo a fini sociali delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità mafiosa. Queste ultime, non solo rappresentano il simbolo della lotta dello Stato contro le organizzazioni criminali nel nostro tessuto economico, ma devono soprattutto sia essere un'opportunità concreta per risollevare l'economia del Paese, sia offrire opportunità di aggregazione sociale, dedicate *in primis* ai nostri giovani. Andranno progettate idee per la creazione di centri sportivi, culturali, di studio e di svago. Solo in questa maniera potremo affrontare e vincere le sfide che la lotta alla criminalità organizzata pone di fronte a noi. Solo così saremo in grado di massimizzare lo straordinario lavoro portato avanti dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura sul piano della repressione. Solo così, infine, vinceremo la battaglia culturale a favore della giustizia e della legalità.

Presidente, per l'Agcom la Grexit è già una realtà conclamata, cioè la Grecia già non è più in Europa, al punto che nel video ufficiale per la fine del *roaming* in Europa, l'Autorità di vigilanza per le telecomunicazioni cancella con un colpo di spugna Atene e tutti i suoi concittadini (lo potete trovare sul canale YouTube di Agcom). A Bruxelles, il breve *spot* suscita subito i malumori del Governo di Alexis Tsipras che manifesta apertamente il suo disappunto

Sull'assunzione di David Nebiolo avevamo già protestato, perché secondo noi non aveva le caratteristiche per occupare quel posto (l'affidamento dell'incarico di comunicatore era avvenuto in qualità di amministratore delegato di un ristorante romano). La questione della sua assunzione in barba alla legge (abbiamo anche fatto un esposto a Cantone, che finora non ha mosso un dito) è rimasta in sospeso. Certo è difficile intervenire in questo momento mettendo in discussione l'operato l'operato di Cardani che in questo momento è l'ago della bilancia nella disputa in corso, molto importante, fra la francese Vivendi e la Mediaset di Silvio Berlusconi. La posta in gioco, signori, è molto alta: Agcom è anche l'autorità che vigila sulla *par condicio* in tempi elettorali e fa quindi il bello e il cattivo tempo nel decidere chi ha sforato e chi no nei passaggi televisivi e creare l'opinione pubblica, soprattutto in un Paese in cui la componente

lo cancelli così come ha cancellato la Grecia dal video. Lo dico perché ci è arrivata appena adesso la comunicazione dell'invito per la relazione annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

I numeri non ci convincono, signora Presidente, non ci convincono la mancanza dei dati numerici e la mancanza di trasparenza di questo Governo. Sottolineo che da oltre due mesi il Ministero non fornisce più i dati sulle presenze nel sistema di accoglienza nel cruscotto giornaliero. Abbiamo dei dati sommari che sono però importanti. Alla fine del mese di dicembre nel sistema di accoglienza si registravano poco più di 176.000 Ebbene, al 18 aprile, ultimo dato disponibile, di presenze ce n'erano poco più di 180.000, 3.000 o 4.000 unità in più come sia possibile questo minimo incremento, tenuto conto che dall'inizio dell'anno sono quasi 70.000 le richieste di asilo pervenute e che i ricollocamenti, quindi i numeri relativi a coloro che vengono mantenuti nel sistema di accoglienza, sono poco più di 2.500. Insomma, noi dovremmo registrare 220.000-230.000 presenze nel sistema di accoglienza. Ci domandiamo dunque perché viene comunicato un numero così basso e ci domandiamo se sono migliaia gli allontanamenti non giustificati dei richiedenti asilo. Ci sta venendo il dubbio che una persona che magari è scappata dalla guerra o da persecuzione, una volta che ha ottenuto lo *status* di rifugiato, di protezione sussidiaria, venga sbattuta immediatamente fuori dal sistema di accoglienza e non venga più tenuta per mesi come veniva fatto in precedenza. Insomma sarebbe grave che chi scappa da guerre e ottiene lo stato di rifugiato, venga sbattuto fuori dal sistema di accoglienza e che invece, nello stesso sistema di accoglienza, vengano mantenuti decine di migliaia di richiedenti asilo che poi si riveleranno dei clandestini. Stiamo ponendo un problema molta serio, signora Presidente, tenuto conto che l'immigrazione fuori controllo da parte di questo Governo comporta dei costi sociali, dal punto di vista della sicurezza, e soprattutto dei costi in termini economici. Il ministro Padoan dice che quest'anno la gestione dell'immigrazione cuba 4,7 miliardi di euro e oltre la metà di questi vengono spesi per l'accoglienza. sollecitiamo nuovamente il Ministro dell'interno perché dia risposta alla nostra interrogazione. Lo prometto qui: d'ora in avanti ogni settimana interverrò sulla mancata risposta alle nostre interrogazioni e ogni due settimane depositeremo una nuova interrogazione, perché venga data risposta risposta non tanto al Gruppo della Lega Nord, ma ai cittadini italiani che meritano da questo Governo la trasparenza che voi state facendo mancare.